Grazie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

Comunico che in data 12 settembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

in Aula per un'informativa. Lo dico senza polemica, ma credo che sia necessario in questa fase avere un chiarimento pubblico e anche alcune delucidazioni sulla nuova piccola piccola ondata di Covid. Abbiamo letto sui giornali informazioni discordanti, quindi possiamo dire che non abbiamo una vera e propria informazione, ma articoli più o meno allarmistici.

ci illustri la situazione epidemiologica rispetto a questa ondata di Covid. Abbiamo visto le circolari di agosto, ma rimane una certa confusione su che cosa fare per i lavoratori e per i pazienti più fragili, soprattutto in una fase come questa, ossia nel pieno dell'inizio dell'anno scolastico.

passare da tutto quello che c'è stato a non parlare più delle infezioni credo sia un errore; invece, comunicare con la popolazione con buon senso, anche rispetto alle procedure che devono tenere i medici di famiglia o i pediatri, aiuterebbe a gestire la fase di normalizzazione della

buon senso. Senza voler fare dell'allarmismo e sapendo che oggi, grazie al cielo e grazie alla scienza, i casi di Covid sono molti ma non gravi, resta un problema importante che riguarda gli anziani e i pazienti fragili. Occorre quindi che il Ministro venga in Parlamento e illustri in maniera puntuale cosa il Governo intende fare fare innanzitutto per una corretta informazione a queste persone, ma soprattutto per la tutela della loro salute. Affronteremo il tema della sanità anche all'interno della legge di bilancio e per noi è la priorità, ma in questo momento, visto anche l'avvio dell'anno scolastico, riteniamo importante tornare sul tema delle vaccinazioni e dare informazioni chiare e certe alle famiglie e, in particolare, ad anziani e pazienti fragili.

voterà con grande convinzione a favore di questo provvedimento. È stato svolto un ottimo lavoro dal Governo anche in Commissione e per questo ringrazio il sottosegretario Bitonci e il relatore Paroli. Il testo ha trovato un'ampia convergenza e mi auguro che questo si riscontrerà nella votazione finale. Trattandosi peraltro di una delega, si fissano dei principi sui quali si continuerà a lavorare. Credo che l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il sistema degli incentivi alle imprese sia condiviso, condiviso, a maggior ragione in questa fase in cui l'armonizzazione degli interventi nazionali e locali e la migliore gestione delle risorse del PNRR consigliano al Paese la coesione. Sottolineo con favore l'erogazione della terza rata e sicuramente arriverà anche la quarta. Connetto questo tema all'altro perché è tutto un insieme di misure che ci devono aiutare ad affrontare al meglio

comune delle forze parlamentari e può rappresentare una pietra miliare per il lavoro dei prossimi anni a sostegno delle imprese. Il termine è di ventiquattro mesi, ma noi ci auguriamo, che il Governo possa agire con una rapidità ancora maggiore viste l'urgenza dei problemi e le questioni importanti che ci impone la competitività dei sistemi economici. Le misure che saranno assunte avranno sicuramente un effetto leva sull'economia nel suo complesso. di un'armonizzazione e di una razionalizzazione del sistema degli incentivi. Anche noi nella nostra esperienza di parlamentari e nel dialogo con il sistema produttivo a volte riscontriamo la farraginosità

sulla gestione di queste risorse sia assolutamente necessario. Abbiamo avuto anche una fase storica in cui il sistema degli incentivi è stato oggetto di numerosi interventi. Nella fase della pandemia, che abbiamo vissuto con grande impegno in Parlamento, è ovvio che si è intervenuti anche con misure temporanee e finalizzate al sostegno di settori che hanno vissuto - direi tutti - una stagione drammatica, senza precedenti, che ha provocato il blocco del Paese. È poi arrivato il tema dell'energia e delle materie prime che costano di più e la vicenda dell'aggressione all'Ucraina ha avuto ed ha incidenze che i vari Governi, e quindi anche il Governo italiano, hanno dovuto affrontare.

Meglio una gestione più razionale, essendo l'orizzonte del 2026 molto vicino. L'attuale Governo sta cercando di non perdere quelle opportunità e quindi, se la scansione temporale, di cui il ministro Fitto ha più volte parlato suggerisce in alcuni casi

quindi, che anche la vicenda della revisione del PNRR e del negoziato che si sta facendo a livello europeo sia strettamente connessa a tutta questa materia che va poi nel suo complesso raccordata. Per Forza Italia bisogna ricomporre la frammentazione degli aiuti e degli incentivi riconducendola a un piano

tutte collegate per affrontare una navigazione che sappiamo essere impegnativa. C'è poi il tema degli aiuti di Stato che sono vietati dall'Unione europea. europea. Noi siamo europeisti e Forza Italia si fa un vanto di questa vocazione, ma l'Europa deve essere realista. Giorni fa i BRICS si sono riuniti, si sono allargati ad altre realtà dell'Africa e dell'Asia, ci sono blocchi continentali come la Cina e l'India che agiscono sui mercati:

dell'armonizzazione degli incentivi, una visione più realistica dei cosiddetti aiuti alle imprese vada affrontata, perché in molti casi dobbiamo difendere i nostri settori produttivi, penso alla trasformazione dell'industria siderurgica, chiamata anche a sfide di sostenibilità, quando in altre parti del mondo producono acciaio inquinando e non non rispettando alcuna legge. Esorto quindi il Governo, anche sotto questo profilo, ad affrontare in piedi un confronto con la realtà europea perché il divieto sugli aiuti di Stato non precluda la possibilità di un incentivo sano e anche la difesa dell'economia europea, non solo italiana, rispetto a una concorrenza

hanno avuto un confronto con le categorie economiche, di cui abbiamo ascoltato le istanze come si fa in un processo di decisione trasparente e responsabile. Il testo del Governo è stato migliorato anche con nostri emendamenti, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, che è un *work in progress*, un lavoro continuo da raccordare con tutti gli altri interventi, anche riflettendo molto su cosa voglia dire oggi aiuto le imprese cosa voglia dire legittima difesa in un mondo in cui ci sono colossi - ho parlato dei BRICS, ma potrei parlare di Amazon, di Google e di altri - che entrano in tutti i settori e non pagano tasse. Questo è un tema che anche in queste ore dovremmo discutere, perché se è giusto chiedere soldi alle banche, a maggior ragione è giusto chiedere soldi a Bezos, a Zuckerberg e a chi accumula guadagni enormi e non paga nulla. *(Applausi)*. Poi l'artigiano con i 1.000 euro di incentivi si deve sentire quasi come un perseguitato dall'umanità. C'è quindi uno squilibrio, ma anche questa è materia che dovremmo regolare altrove. Ho visto che anche il vice ministro Leo ha annunciato l'anticipazione di misure in quel campo che l'Europa tarda ad ad assumere. In conclusione, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento, esortando il Governo a esercitare, nei tempi più rapidi possibili, questa delega che aiuterà molto il nostro sistema produttivo.

il provvedimento che esaminiamo oggi è solo l'ultimo in ordine di tempo che si va ad aggiungere ad altri tasselli fondamentali che questo Parlamento ha realizzato insieme al Governo negli ultimi mesi in tema di impresa, semplificazione e crescita. Un provvedimento orgogliosamente e ampiamente condiviso. In soli dieci mesi di buon governo del centrodestra abbiamo approvato numerose misure per favorire la crescita delle imprese e la competitività del comparto industriale italiano. Dunque, questo provvedimento costituisce un ulteriore passo di rilievo a cui ne seguiranno ben presto altri, lungo quel percorso già tracciato che riteniamo possa assicurare sviluppo al Paese: vedasi il cosiddetto decreto *asset* e il cosiddetto decreto TIM sugli investimenti di interesse strategico, entrambi già all'esame all'esame di questo ramo del Parlamento. Penso a loro in particolare e al tema dell'accesso al credito per le imprese, o ai problemi legati ai ritardati pagamenti dei lavori eseguiti in favore della pubblica amministrazione, oppure ai tanti crediti fiscali ancora incagliati a causa degli scellerati *bonus* distribuiti a pioggia. Ma penso anche all'eccessiva pressione fiscale che grava ancora su quelle imprese che vogliono investire, in particolare in innovazione, un settore che merita di essere accelerato e tutelato, perché *startup* e innovazioni tecnologiche rappresentano oggi un'importante fetta del nostro PIL nazionale. D'altronde, sono i dati e le statistiche che lo certificano, come dirò più avanti. Su questi tre filoni auspico che il Governo lavori intensamente nei prossimi mesi per fornire risposte concrete ai cittadini e a tutte quelle imprese che non vogliono smettere di lottare contro la crisi e credono seriamente di poter continuare a investire nella nostra Nazione. Per fare questo, però, dobbiamo garantire loro un quadro di maggiori certezze che favorisca e non certo penalizzi gli imprenditori, proseguendo nella scia della sburocratizzazione, eliminando lacci e lacciuoli che da troppo tempo attanagliano le nostre imprese. Voglio ora brevemente mettere in luce alcuni degli aspetti positivi del provvedimento che stiamo esaminando. Questo disegno di legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché di semplificazione delle relative procedure, punta anzitutto a ridisegnare la cornice di regole in questa materia, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo. Per la prima volta dopo tanti anni - va detto - questo Governo di centrodestra e tutta la maggioranza che lo sostiene, di cui orgogliosamente facciamo parte, si è posto l'obiettivo ambizioso di razionalizzare il complesso delle norme vigenti in tema di agevolazioni alle imprese, per garantire così una migliore pianificazione ed attuazione. Basti pensare che l'attuale quadro normativo è frastagliato in quasi 2.000 incentivi nazionali e regionali non sempre tra loro coerenti; ad esempio, nel 2021, si sono registrati 1.982 interventi agevolativi, di cui 229 di matrice nazionale e 1.753 regionali, affidati alla gestione di ben 643 soggetti concedenti: numeri pazzeschi, da capogiro. Serviva dunque un riordino, una semplificazione fatta di poche e semplici regole chiare e certe, così come di princìpi trasparenti: un intervento resosi più che mai necessario proprio per delineare metodi e criteri di definizione degli incentivi, affinché questi stessi siano realmente in grado di attrarre e stimolare investimenti nuovi e innovativi e possano spingere il sistema produttivo verso frontiere tecnologiche più avanzate, assicurando un supporto a tutte le fasi di sviluppo di un'impresa e a specifici obiettivi, a partire da quelli legati alla transizione verde, alla salute, alla coesione sociale, economica e territoriale. Da un sistema di incentivi ben congegnati, infatti, un sistema che tenga conto delle potenziali sinergie tra gli interventi e che riesca a prevenire eventuali reciproci spiazzamenti e sovrapposizioni può dipendere la competitività del sistema produttivo italiano e la sua capacità di trainare l'economia e la crescita del Paese, garantendo al tempo stesso l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica; la capacità, quindi, di poter offrire un quadro netto e preciso ad eventuali investitori che vogliano venire ad investire in Italia. Ringrazio ancora il Governo per aver dimostrato sensibilità su questi temi, che abbiamo posto sin da subito come prioritari: primo, la valorizzazione del contributo all'imprenditoria femminile; secondo, la piena di equiparazione tra professionisti e imprese al fine di accedere ad agevolazioni ed incentivi; terzo, l'attenzione all'industria del turismo, che - ricordo - da sola vale per l'Italia oltre il 13 per cento del PIL, affinché possa anch'essa usufruire delle agevolazioni in materia di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, cosa finora di fatto preclusa. Da ultimo, signor Presidente, ma non per questo meno importante, vi è l'attenzione verso un settore, quello dell'innovazione tecnologica, che è un futuro già presente, che può dare milioni di posti di lavoro ai nostri giovani e favorire il rientro dall'estero, dove si investe costantemente sul sistema delle *startup* a strascico. Mi lasci solo sottolineare, signor Presidente, che l'ecosistema dell'innovazione italiano, seppur in netta crescita, muove purtroppo volumi ancora distanti da quelli presenti in altri Paesi europei, con dimensioni economiche similari o inferiori, ed ha una grande necessità di sostegno da parte delle istituzioni tutte per provare a recuperare quel divario purtroppo ancora esistente. Per quanto riguarda il raffronto con altri Paesi, basti pensare che nel 2022 (anno record in Italia) sono stati investiti circa un miliardo e 800 milioni verso le *startup* e le imprese innovative; un dato che può sembrare interessante, ma che diventa poco rilevante se paragonato ai 6 miliardi investiti in Spagna, agli 11 miliardi investiti in Francia e ai 15 addirittura in Germania. Uno dei motivi di questo ritardo è il modo in cui spesso si guarda alle *startup* e alle piccole e medie imprese innovative, considerate come delle imprese di ragazzi e per ragazzi. Invece è evidente il loro contributo fondamentale non solo al rilancio economico di un Paese, ma soprattutto al suo sviluppo in termini di imprenditoria veloce, *smart* ed efficiente, al funzionamento agevolato del mondo nuovo che ci aspetta. Nonostante gli alti e bassi, l'ecosistema italiano dell'innovazione sta attraversando una fase di crescita. Ci sono le basi per essere il prossimo potenziale centro di attrazione per molti operatori internazionali, soprattutto a Sud, grazie alle ZES, come dimostrato da una crescita del 48 per cento del mercato del nostro Paese, anno su anno (2021-2022), crescita che assume ancor più valore se confrontata con quella del 6 per cento del mercato francese e con le crescite negative di Spagna e Germania. Condividiamo la *ratio* di fondo di reimpostare il sistema degli incentivi, definendo pochi e semplici strumenti fiscali e finanziari, tali da poter essere adattati alle diverse e specifiche strategie, che possono evolvere e cambiare nel tempo. In tal senso, abbiamo ben chiara la strategia da seguire da qui innanzi: realizzare un contesto più competitivo per le imprese e più attrattivo nei confronti

con l'affiancamento di altri provvedimenti che contiamo di poter mettere in cantiere, in un clima di continua collaborazione tra Parlamento e Governo, in questo difficile momento economico e sociale, anche mettendo in campo la creatività italiana. Abbiamo iniziato un percorso e lo dobbiamo portare avanti nell'interesse del sistema Paese. Il monito che credo sia il più importante e che ciascuno di noi dovrebbe rammentare è solo uno: tornare a crescere per far tornare grande l'Italia. Continueremo ad affiancare e a supportare questo Governo, per rendere ancor più concreta la politica che sta portando avanti, fatta di meno tasse e più interventi a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Siamo convinti che il Paese o, per meglio dire, la squadra Italia potrà reagire; e ce la farà se ognuno, a cominciare da noi stessi, farà fino in fondo la sua parte. Noi continueremo a fare la nostra: continueremo ad investire per il futuro di questa Nazione. È per questo motivo che il nostro Gruppo voterà a favore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ognuno di noi, quando decide come votare un provvedimento, parta dal considerare qual è l'ambizione del provvedimento stesso. Questo provvedimento nasce con l'ambizione di riordinare la materia degli incentivi alle imprese;

di cui 229 dallo Stato e 1.753 dalle Regioni, per un ammontare significativo di 146 miliardi. Ovviamente questi 146 miliardi pesano sul terreno dell'economia, in termini di agevolazioni concesse per la crescita produttiva. L'esigenza di fare ordine, di stabilire delle e di coordinare l'attività dello Stato centrale e delle Regioni e, nello stesso tempo, l'esigenza di evitare che i finanziamenti siano frammentati in strumenti che moltiplichino i soggetti che gestiscono

lo spirito, l'impostazione, la necessità e anche lo sforzo che la Commissione ha fatto, però l'obiettivo è raggiunto molto parzialmente,

aiutarle in quella direzione, in particolare il tessuto delle piccole e medie imprese che rappresentano la forza produttiva del nostro Paese.

uscita dalle fonti e dai settori tradizionali. Pensiamo a un settore strategico come quello energetico, di cui tutti noi in questi mesi discutiamo: quante volte abbiamo discusso anche della crisi energetica? Sappiamo tutti

mi corre l'obbligo di ringraziare il sottosegretario Bitonci, il presidente Luca De Carlo e il relatore Adriano Paroli per l'attenzione che hanno prestato alle opposizioni e in particolare agli emendamenti provenienti dal mio Gruppo.

l'Italia ha una storica tradizione industriale e, nonostante la complessità del Paese, continua ad averla,

con talmente tanti balzelli che è difficile arrivare al traguardo. Eppure ci riusciamo, ci riescono le nostre imprese e il nostro tessuto imprenditoriale. Chi parla viene da Torino, che era conosciuta come la città della grande fabbrica. Oggi non lo è più, quella grande fabbrica purtroppo non ha la stessa rilevanza nel Paese e nella mia città, ma ne abbiamo altre, perché nel frattempo l'economia è cambiata e la *green economy* è entrata nel linguaggio dei giovani imprenditori. Molti mi scrivono raccontandomi di *startup* fantastiche, che nel giro di poco tempo vengono inserite nell'elenco delle grandi innovazioni a livello mondiale. Dico questo, che sembra non c'entrare con l'argomento è molto vero che serve un riordino di tutta la parte degli incentivi e credo che anche il prossimo Parlamento europeo debba rivedere la normativa sugli aiuti di Stato. Lo dico da europeista convinta, ma in questi anni è sembrato che l'Europa avesse paura delle sue imprese, che nutrisse una ideologia astratta verso la concorrenza e che fosse talmente tanto concentrata sugli aiuti di Stato alle imprese europee da non accorgersi dell'arrivo dei finanziamenti e dei grandi *buyer* stranieri, cinesi, indiani e di altre nazioni, che di fatto hanno spolpato il sistema industriale europeo. Quindi mi auguro che si riveda tutto il sistema degli aiuti da aiuti da dare al nostro sistema produttivo, per evitare che evapori completamente. Parto da questo principio, perché i provvedimenti si devono parlare tra di loro. Questo è un provvedimento che va verso una direzione,

prima lo cambiamo e poi facciamo la norma sugli extraprofitti *(Applausi)*. Se facciamo prima la norma sugli extraprofitti bancari in un sistema che finanzia le imprese attraverso le banche, temo che abbiamo fatto un danno alla nostra economia.

non si ha una visione di sistema industriale nel nostro Paese. L'ultima è stata quella di Industria 4.0, che però - lo dico,

perché capisce, avendo avuto anche altre funzioni governative in passato,

dico sempre, quando i Paesi emergenti diventano finalmente ricchi, chiedono *made in Italy*, per cui vuol dire che la nostra industria, la nostra impresa e la nostra bellezza arrivano subito.

Signor Presidente, colleghi e membri del Governo, anticipo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Ringrazio il Presidente della 9ª Commissione per aver permesso che il lavoro emendativo, frutto delle varie sensibilità politiche, potesse alla fine esprimere un documento che, per stessa ammissione del Governo, è quanto meno migliore della sua forma originale. Noi abbiamo quindi condiviso buona parte dei principi posti in essere e di alcune misure possiamo ritenerci soddisfatti, come nel caso dell'equiparazione dei professionisti alle piccole imprese nell'accesso agli incentivi, così come richiesto dalla normativa europea; oppure, come nel caso dell'emendamento del MoVimento 5 Stelle, sul rinnovo del DURC per le imprese quindici giorni prima della scadenza: misura richiesta da anni dalle associazioni di categoria e finalmente attuata. Molti sono i punti su cui avremmo certamente preferito maggiore approfondimento e attenzione del Governo. Non mi dilungherò su quanto i miei colleghi hanno già evidenziato in discussione generale, ma certamente il *click day*, la perequazione strutturale nelle aree depresse e la differenziazione di genere nell'accesso agli incentivi rientrano in questo monito. Né è passato inosservato l'emendamento del relatore che ha messo in dubbio la presenza degli incentivi fiscali nel codice da elaborare; né tantomeno l'uso strumentale delle inammissibilità con cui alcuni importanti emendamenti sono stati cancellati. di questo provvedimento, signor Presidente, perché riteniamo prioritaria la funzione di tale testo, la cui finalità è la necessità di rimuovere gli ostacoli che limitano l'efficacia delle politiche di incentivazione per le imprese, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione. In questo contesto, va segnalato che Banca d'Italia ha depositato una memoria che compie un'analisi storico economica sull'attuazione in Italia di politica industriale dal periodo prepandemico ad oggi, soffermandosi sull'importanza della costruzione progressiva di un sistema di aiuti finalizzati al sostegno del tessuto produttivo italiano ed evidenziando un certo grado di inefficienza nella allocazione delle risorse pubbliche, se rapportata con la media degli altri Paesi europei, sottolineando l'importanza della stabilità e della certezza delle normative sull'incentivazione. Soprattutto, aggiungo che bisogna lavorare per eliminare il divario esistente tra Centro Nord e Mezzogiorno sulla capacità di investimento. di misure concrete, che necessitano inevitabilmente di una lungimiranza, che sembra però difficilmente rintracciabile nell'azione e nei provvedimenti di questo Governo. Mi riferisco al poco coraggio dimostrato nel non accogliere gli emendamenti che chiedevano l'esplicita eliminazione dei SAD, i sussidi ambientalmente dannosi. Signor Presidente, è ben chiaro a tutti e noi non dimentichiamo che questo provvedimento è una legge delega, che rappresenta un piccolo passo avanti, viste le misure che contiene. Come ho detto all'inizio, noi voteremo a favore di questo disegno di legge, del quale abbiamo condiviso alcuni contenuti, apportando importanti modifiche.

Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, scriveva il conte Carlo Dossi che lo scopo della burocrazia è condurre gli affari dello Stato nel peggior modo possibile e nel più lungo tempo possibile. Quel che Dossi ai suoi tempi non poteva prevedere né tantomeno immaginare è che la burocrazia non avrebbe distrutto solo l'amministrazione dello Stato, ma avrebbe anche esteso il suo potere velenoso agli affari privati.

Risulta quindi inutile aggiungere come sia evidente che più di qualche cosa non abbia funzionato. Oggi siamo qui proprio per scrivere una nuova fase del rapporto tra Stato e imprese. Scopo di questo provvedimento è, infatti, la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere tutti quegli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Abbiamo quindi individuato una serie di obiettivi fondamentali di questa riforma. Tra i più importanti: razionalizzare l'offerta di incentivi ordinando dei modelli di agevolazioni; armonizzare la disciplina di carattere generale coordinandola in un unico testo normativo, il cosiddetto codice degli incentivi; programmare degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti; garantire l'agevole conoscibilità delle misure di incentivazione da parte degli imprenditori in relazione agli obiettivi e alle condizioni; digitalizzazione e semplicità delle procedure, al fine di ridurre nella misura più ampia possibile gli oneri burocratici a carico degli imprenditori; un'ampia coesione sociale, economica e territoriale con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale del Paese. È un provvedimento, questo, a cui la 9a Commissione del Senato ha lavorato a lungo e mi unisco ai ringraziamenti fatti ieri dal collega Bergesio al nostro Presidente della Commissione affinché si ottenessero delle migliorie. Di particolare rilievo è quella, fortemente voluta dalla Lega, che stabilisce ai fini dell'accesso agli incentivi di fatto un principio di equiparazione tra professionisti e imprenditori. Sì, finalmente siamo stati capaci di far cadere quel muro che separava, ai fini delle incentivazioni, professionisti ed imprese, e verranno così garantite pari opportunità eliminando quelle disparità di trattamento che per anni hanno impedito un organico sviluppo delle libere professioni in Italia. In base alla formulazione che esce dalla Commissione, il processo di revisione sarà capace di puntare alla ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle agevolazioni, quali: il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale; nonché la facilitazione nell'accesso nell'accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione o altri ambiti e finalità del sostegno. La storia degli ultimi decenni d'Italia lascia ben intendere che i problemi economici di un Paese non si risolvono per niente con l'elemosina di Stato o con gli aiuti a pioggia o con la demonizzazione della ricchezza. Una delle differenze fondamentali tra destra e sinistra sta proprio nel fatto che la sinistra ritiene che lo sviluppo dell'economia sia un compito dello Stato. Noi riteniamo che tale azione spetti alle imprese e che lo Stato debba essere d'aiuto a queste, affinché realizzino tale obiettivo. Un Paese che intende risollevarsi e percorrere con risolutezza virtuosi sentieri di crescita deve rimettere al centro della scena la figura dell'impresa, che sa coniugare il proprio bene con il bene comune. Gli imprenditori italiani negli ultimi anni hanno vissuto uno dei momenti più bassi in quanto a reputazione e considerazione del loro ruolo nel consesso sociale. Il retaggio culturale imposto dalla sinistra e tutte le sue sfumature di rosso hanno etichettato chiunque abbia voluto e voglia fare impresa in Italia come un signore che sfrutta i dipendenti, inquina l'ambiente, non paga le tasse e persegue solo il proprio tornaconto a discapito di tutti gli altri. L'eccesso di burocrazia è proprio figlio della presunzione di colpevolezza che le distorsioni del pensiero della sinistra hanno sempre attribuito a chi fa impresa, grande o piccola che sia. Il mutamento culturale che la sinistra ha imposto negli anni ha portato anche ad amplificare tutti quei fenomeni di male affare esplosi negli anni recenti, recenti, che per certi versi sono fisiologici in qualsiasi sistema socioeconomico, e nessuno strumentalizzi o interpreti in modo falsato questa mia affermazione. La sinistra ha fatto in modo di portare questi esempi negativi come prova del loro assunto. L'imprenditore mira esclusivamente a esercitare una funzione utilitaristica di arricchimento personale e questa è una follia. Noi invece, come Governo e maggioranza, crediamo che il fine generale dell'impresa sia concorrere per molteplici vie alla promozione della persona umana e che il reddito sia non il fine esclusivo dell'impresa, ma una parte del sistema dei valori della dinamica economica. L'impresa è la molecola dello sviluppo ed è fatta di individui che prendono in mano il proprio destino senza delegarlo ad altri. Con questo provvedimento - ma non solo - intendiamo valorizzare a pieno le potenzialità del tessuto imprenditoriale, in particolare quello delle piccole e medie, capace di generare sviluppo umano, crescita sociale e di perseguire attraverso la molla del profitto, non fine a se stesso, il bene comune e, quindi, il bene del nostro meraviglioso Paese. Morire sani, ma di fame, non rientra negli obiettivi che questo Governo vuole dare alle imprese e neanche vivere di crocchette di Stato come tanti animali domestici, sempre che fosse possibile. Lo scopo ultimo del segnale inviato è quello di far sentire apprezzata e valorizzata l'azione di centinaia di migliaia di imprenditori che finora hanno operato in un contesto culturale ostile e che ha provocato, come naturale conseguenza, l'asfissiante attenzione dello Stato attraverso controlli severi di molti suoi apparati; controllo che, con estrema ironia della sorte, quasi mai è stato in grado di fermare chi agiva in malafede o addirittura da fuorilegge più o meno organizzato. Finalmente però siamo al cambio di passo: riformare e soprattutto agevolare il mondo degli incentivi alle imprese significa affermare che il Governo c'è e crede in loro; significa dare un messaggio positivo e di coraggio alle nuove generazioni; significa che l'Italia ha un futuro. L'Italia è il Paese che amo: fu questa la dichiarazione d'amore che Berlusconi regalò al nostro Paese per sintetizzare una visione nuova anche per la politica industriale italiana. Sì, perché questa maggioranza ha un obiettivo ambizioso, quasi folle secondo qualcuno: tornare ad avere una politica industriale. Politica e industria: due parole che negli ultimi anni erano diventate antitetiche per la miopia della politica economica della sinistra. Proprio per questo oggi abbiamo il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'istruzione e del merito. Finalmente il centrodestra è unito e ha la forza nuova per ridare quella dignità che la sinistra sinistra ha mortificato in tutti questi anni a chi vuole rendere questo Paese più bello, più forte, più produttivo e innovativo. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito

infatti a incidere sulla capacità competitiva, sull'attrattività delle imprese, sull'indirizzo delle scelte industriali in chiave interna e soprattutto per quel che riguarda il rapporto con le altre economie. Io provengo da una terra come il Veneto e so quanto innovazione, creatività e capacità di resilienza siano da sempre i tratti migliori della piccola e media impresa italiana. Sono le qualità che hanno permesso di avere un ruolo decisivo negli anni della ricostruzione, nello straordinario periodo del *boom*, tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà degli Sessanta, e naturalmente nei decenni successivi fino a conquistare posti di primissimo piano nei mercati internazionali. Questa è quindi una grande storia che è anche presente nonostante tutte le difficoltà attuali e che di certo ha anche un futuro. Le migliori qualità di chi fa impresa sono sempre le stesse; sono quelle che già Luigi Einaudi sottolineava dicendo che migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo fare per molestarli, molestarli, per incepparli e scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge. Sono parole che raccontano benissimo la passione, l'impegno, le ansie e le speranze di chi nel nel proprio lavoro ci mette davvero l'anima, di chi nel proprio lavoro mette tutto sé stesso, di chi crede fino in fondo nella propria attività e trasmette tutto questo ai suoi collaboratori e ai suoi dipendenti. A noi, oggi, soprattutto dentro una crisi che, tra pandemia e guerra in Ucraina, dura ormai da tre anni e mezzo, spetta un compito cruciale: non solo evitare di molestare, inceppare e scoraggiare, ma anche sostenere e promuovere l'attività delle imprese italiane. In questo senso, il tema della revisione del sistema degli incentivi si pone ormai nel dibattito politico da parecchio tempo. È un'esigenza condivisa sia a livello istituzionale che tra le parti sociali, in particolare in questa fase, nel pieno dei processi di transizione in atto con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione, con l'intelligenza artificiale, con la ecologizzazione delle produzioni. Il disegno di legge dovrebbe affrontare tutto questo, è un collegato alla manovra di bilancio e ha nel PNRR la sua genesi. Proprio riguardo al PNRR, non posso però in quest'Aula fare a meno di cogliere come questa occasione, che è decisiva per il sistema produttivo oltre che per tutto il nostro Paese, rischia di essere sprecata. Devo farlo con consapevolezza e con preoccupazione, di fronte ai ritardi, alla scarsa trasparenza e ai troppi miliardi che rischiano di essere persi e di finire nel cestino, soprattutto di fronte all'evidenza di un Governo che sul PNRR ha un problema che è soprattutto culturale, perché fin dall'origine non lo ha condiviso e continua a vederlo come un obbligo, come un fastidio e non come una straordinaria e irripetibile opportunità. A lanciare questo allarme siamo non solo noi, A lanciare questo allarme siamo non solo noi, non solo l'opposizione, ma è tutto il mondo economico e sono anche quelle realtà alle quali si rivolge il disegno di legge. Il provvedimento - come è stato ricordato anche da altri colleghi che sono intervenuti nella sua versione originaria presentava numerosi aspetti critici e noi abbiamo cercato di migliorarlo con delle proposte di modifica. Voglio qui ricordare il principio per cui bisogna assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e alla trasparenza delle procedure, la strategicità dell'interesse nazionale; l'obiettivo di razionalizzare gli incentivi, lasciando però alle Regioni autonomia nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati; la ricognizione e la sistematizzazione delle misure di incentivazione; l'attenzione alla crescita dimensionale, all'aggregazione delle imprese; il rispetto dei tempi e delle attività istruttorie che sono fondamentali per consentire alle imprese la propria programmazione e infine il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria più rappresentative. Tuttavia, rimane una serie di criticità. Come emerso anche nel dibattito in Commissione, la delega fiscale che abbiamo recentemente approvato rischia di sovrapporsi e ingenerare problemi con quanto previsto da questo disegno di legge, in quanto tra i princìpi di delega anche lì sono previsti la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese. Il tentativo da parte del relatore, che pure ringrazio per il lavoro, e del Sottosegretario, che ha seguito con attenzione questo percorso, di stabilire un confine tra le due discipline a nostro avviso non risolve la questione e rimane oggettivamente sullo sfondo il potenziale conflitto tra le due amministrazioni capofila delle due deleghe, e cioè quella che fa riferimento al MEF, ovviamente, e quella del Ministero delle imprese. Non solo, ma avevamo proposto una ulteriore modifica agli interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per la riduzione dei divari territoriali; così come avevamo previsto una serie di misure per favorire la sostenibilità economica delle imprese nel processo di transizione energetica e climatica. Anche sulla parità di genere, che pure è presente come finalità connessa a sostegno dell'imprenditoria femminile, noi

che mi auguro possono essere risolte più avanti: mi riferisco ai limiti del *click day* o soprattutto all'esigenza di valorizzare la potenzialità delle trasformazioni digitali e soprattutto di sostenere le nostre imprese nella penetrazione nei mercati esteri. Qui davvero ritorniamo al limite grande di questo Governo, per cui anche una delega come questa, che contiene alcuni princìpi importanti, rischia di non essere efficace. Affrontare una delega di tale portata senza accompagnarla ad una visione a una strategia compiuta non dà il necessario impulso al rilancio del sistema delle imprese. Servirebbe davvero una politica industriale che questo Governo sta dimostrando di non avere. È il punto centrale della nostra critica: una delega che si pone alcuni princìpi giusti, ma una politica industriale del Governo del tutto assente e lo abbiamo visto nel corso di questi mesi nei molti casi che sono stati affrontati. Per queste ragioni oggi il nostro sarà un voto di astensione, anche in considerazione dei miglioramenti che ci sono stati, favoriti da una convergenza parlamentare, dal momento che stavamo discutendo di una delega, e cioè di norme e principi, ed anche in considerazione del fatto che sono stati oggettivamente prodotti dei miglioramenti. Nei prossimi mesi vigileremo sull'attuazione della delega, sulle risorse complessive, sugli effetti della distribuzione territoriale e settoriale, sugli aiuti alla transizione e saranno questi davvero i punti su cui vedremo se i decreti attuativi saranno capaci di offrire delle risposte. Noi naturalmente saremo pronti al confronto e saremo pronti a lavorare per migliorare ogni misura che verrà presentata, com'è stato in questa occasione. Naturalmente faremo questo se sceglierete finalmente di concentrarvi sui problemi veri del Paese e degli italiani; se vi preoccuperete di come sostenere le nostre imprese, di come far ripartire la nostra economia, di come ridurre divari e diseguaglianze di genere e territoriali e di come portare pienamente l'Italia sulla strada dell'innovazione dal punto di vista climatico e digitale. Ecco, se farete questo, noi continueremo a esercitare quella responsabilità che da sempre ci appartiene. Mi permetto di avanzare qualche dubbio, perché fino a questo momento non lo avete fatto. In questo momento tempo da perdere non ce n'è più e l'Italia ha bisogno di riprendere a crescere in modo equo,

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione riveste indubbiamente una grande valenza, perché ha il grande merito di affrontare una tematica di scottante attualità e di grande importanza, quale certamente è il sistema degli incentivi alle imprese, all'interno di un contesto temporale molto delicato, quale quello attuale; un contesto *post* pandemico che ha messo a dura prova la nostra economia, con le refluenze della guerra russo-ucraina, che hanno determinato un aumento enorme del costo dell'energia e delle materie prime, che il Governo Meloni ha affrontato con grande determinazione e con altrettanto pragmatismo, se è vero com'è vero che a poche settimane dal suo insediamento, all'interno della legge di bilancio 2023, ha stanziato 21 miliardi di euro su 35 complessivi, complessivi, cosa mai accaduta all'interno del nostro contesto nazionale. Nonostante questo, la nostra economia sta andando bene e tutti gli indicatori macroeconomici lo confermano: il PIL nel 2023 registrerà un incremento dello 0,9 con una percentuale superiore rispetto alla media europea, cosa che non accadeva all'interno della nostra Nazione da qualche decennio. Ma il sistema delle imprese in Italia deve convivere

con l'aumento dei tassi di interesse che la BCE ha stabilito per combattere l'inflazione, che determina problemi aggiuntivi soprattutto per le imprese sottocapitalizzate che - come tutte le statistiche confermano - insistono all'interno di contesti territoriali ubicati nel Mezzogiorno della nostra Nazione. Nazione. Ecco perché il sistema degli incentivi alle imprese riveste un'importanza assolutamente strategica, laddove la partecipazione a bandi per ottenere contributi a fondo perduto o a tasso agevolato e per ottenere crediti di imposta rappresenta talvolta l'unica strada possibile, per le nostre imprese, per migliorare la capacità produttiva e per rimanere all'interno del mercato, cioè all'interno di un contesto temporale di competizione globale, un contesto in cui le nostre imprese devono competere con altre imprese che, all'interno dei rispettivi territori, registrano una pressione fiscale e tributaria nettamente inferiore e un costo del lavoro nettamente inferiore del lavoro nettamente inferiore - mi riferisco ovviamente alle imprese asiatiche, laddove le norme sono molto meno stringenti sul tema del rispetto ambientale - perché sostengono costi di produzione nettamente inferiori. Ecco perché questo disegno di legge è molto importante. Esso si pone l'obiettivo di semplificare, di determinare una programmazione degli interventi assolutamente capillare e di coordinare tutti gli strumenti per evitare le duplicazioni. Il Il panorama nazionale degli incentivi alle imprese comprende un universo assolutamente eterogeneo, la cui complessità è stata incrementata negli ultimi anni anche per

secondo la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, dove vengono monitorati tutti i tipi di aiuti di Stato ad eccezione di quelli che insistono all'interno del comparto agricolo e della pesca - nel 2021 sono stati 1.987 gli interventi di sostegno, di cui 1.638 gestiti dalle amministrazioni regionali e 198 dalle amministrazioni centrali dello Stato. Sono stati 643 i soggetti concedenti, che hanno determinato delle agevolazioni per 146 miliardi di euro, con 314 miliardi di euro di investimenti attivati in maniera complessiva.

anche come risposta alla crisi pandemica. E credo che essi siano assolutamente indicativi e testimonino l'assoluta necessità di un intervento normativo, che è stato presentato al Parlamento e che può davvero determinare una semplificazione del quadro e un coordinamento di tutti questi strumenti, per evitare delle duplicazioni.

Paroli e al contributo di tutti i commissari, che hanno cercato di presentare emendamenti migliorativi del testo, che sono stati in alcuni casi approvati (sia della maggioranza che dell'opposizione). Basti pensare anche all'articolo 1, all'interno del quale sono stati inclusi, nell'ambito della delega al Governo, anche gli incentivi di carattere fiscale, che credo abbiano rappresentato una importante modifica al testo inizialmente predisposto. sono assolutamente condivisibili i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega. Mi riferisco alla stabilità nel tempo e all'adeguatezza, alla programmazione degli interventi, alla chiarezza, alla digitalizzazione, all'uniformità delle procedure, con una particolare attenzione - come è stato evidenziato anche da chi mi ha preceduto - all'imprenditoria femminile, alla imprenditoria giovanile, ai professionisti che possono accedere anche al sistema degli incentivi con particolari premialità che sono state immaginate per quanti si prendono l'impegno di assumere soggetti disabili. Per questo credo che questo testo sia assolutamente importante.

anche attraverso l'implementazione di soluzioni tecniche per superare il fenomeno del *click day* nelle assegnazioni degli incentivi, che ritengo in una fase pandemica abbia rappresentato probabilmente l'unica soluzione possibile in tempi brevi per dare sostegno alle imprese, ma certamente non

e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) per il rilascio accelerato delle certificazioni, al fine di determinare uno snellimento delle pratiche burocratiche amministrative, che troppo spesso rappresentano un ostacolo a percorsi

delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

il disegno di legge n. 727 reca disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Il provvedimento, trasmesso dalla Camera dei deputati, assunto quale testo base dalla Commissione, non è stato oggetto di modifiche nel corso della trattazione in sede redigente, conclusasi con il mandato unanime a riferire favorevolmente. L'articolo 1 del disegno di legge demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica, da avviare a decorrere dall'anno 2024, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Tale *screening* è finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e a rallentare la progressione della malattia, mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che a ottenere diagnosi precoci della celiachia. Si prevede che lo schema del citato decreto sia sottoposto a una serie di pareri, tra cui quello delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, si autorizza per l'attuazione del citato programma pluriennale una spesa pari a 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, al quale è affidato il compito di studiare ed elaborare le risultanze dello *screening* in oggetto e pubblicare annualmente una relazione sul sito Internet istituzionale del Ministero della salute. Si prevede che i 13 membri dell'osservatorio durino in carica tre anni e che il loro incarico possa essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita. L'articolo 3 prevede campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale ad opera del Ministero della salute, con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del suddetto programma di *screening*, autorizzando a tal fine la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dal 2024. Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

per rappresentare innanzitutto la volontà pressoché unanime della Camera dei deputati rispetto al provvedimento in esame, che è stato licenziato - se non ricordo male

che, come recita l'articolo 32 della nostra Costituzione, devono essere curati in maniera omogenea dal Nord al Centro e al Sud, al netto del censo e della provenienza geografica, in coerenza

che si inserisce all'interno del novero della cosiddetta prevenzione, che è fondamentale in questo momento storico per il nostro sistema sanitario nazionale. Voglio ricordare a tutti che, insieme a una maggiore dotazione del Fondo sanitario nazionale, servono sicuramente nuovi modelli organizzativi, ma anche la cosiddetta prevenzione. Prevenire porta a diagnosticare prima le patologie, a non farle conclamare, a curare opportunamente i cittadini italiani e, come effetto secondario, a far risparmiare le casse del fondo sanitario nazionale.

Signor Presidente, colleghi, oggi l'Assemblea del Senato esamina un testo legislativo che introduce importanti disposizioni normative riguardanti la vita delle persone, prestando in modo particolare la giusta attenzione all'importanza di una diagnosi precoce per il diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Per quanto riguarda la celiachia, se vogliamo citare qualche dato, si tratta di una malattia fortemente sottostimata in Italia: sono circa 233.000 i celiaci. Attenzione, però, perché solo il 40 per cento dei pazienti ha ricevuto una diagnosi e può, di riflesso, accedere alle cure. Si stima che ci siano infatti altre 400.000 persone che, al contrario, non hanno ricevuto una diagnosi corretta. Lo stesso vale per il diabete di tipo 1.

1. Come si evince dai dati Istat, questa patologia colpisce lo 0,5 per cento della nostra popolazione. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, l'esordio della malattia è avvenuto proprio nell'età evolutiva. Il 10 per 20.000 pazienti - ha un'età inferiore ai diciotto anni. Vale la pena ricordare quanto sia cruciale diagnosticare in maniera precoce questo tipo di patologia. È questo lo spirito della legge che ci accingiamo ad approvare oggi, perché il nostro nemico tende purtroppo - e spesso

che, se non trattata adeguatamente, predispone a diverse complicanze, che possono compromettere gli organi vitali. Basta pensare ai malati che, se non precocemente diagnosticati e adeguatamente curati, rischiano di sviluppare una forma di chetoacidosi diabetica fino ad arrivare all'edema cerebrale e purtroppo al coma. Per questo, sia nel caso della celiachia sia in quello del diabete di tipo 1, la diagnosi precoce è una forma di prevenzione importante e fondamentale. Com'è noto, il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera, oggi qui presentato al Senato anche dal sottoscritto e dalla collega senatrice Sbrollini, ha come obiettivo, comune a tutti i testi di legge in materia, di prevenire i danni causati dall'evolversi della malattia, che potrebbero essere limitati,

pediatrica, dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra uno e diciassette anni, a partire appunto dal 2024. Grazie a questo *screening* sarà infatti possibile individuare gli anticorpi e rallentare l'evoluzione di queste due malattie. La rivoluzione degli *screening*, al di là delle specifiche patologie, rappresenta davvero una svolta nella prevenzione, che è fondamentale. Tante volte, questa è l'unica forma di controllo di patologie che, nel momento in cui si cronicizzano, tendono ad assumere la forma di patologie multiorgano, che coinvolgono cioè più organi, con costi enormi per le famiglie oltre che per il Servizio sanitario nazionale.

Questo provvedimento, com'è noto, fa seguito a quanto già previsto nella scorsa legge bilancio, in cui è stato istituito un apposito fondo allo scopo di finanziare futuri investimenti normativi per la realizzazione del programma di *screening* che questa legge rifinanzia, come ho appena accennato, con importanti e significative risorse). L'osservatorio nazionale sul diabete e sulla celiachia analizzerà i risultati del programma di *screening* sopracitato. Un altro aspetto importante è quello dell'informazione. Il disegno di legge, infatti, prevede la promozione di campagne periodiche di sensibilizzazione sociale proprio sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica: informare, sensibilizzare e formare. Come abbiamo infatti visto dai dati, sono tanti, troppi, troppi, i casi sommersi. Occorre per questo che istituzioni, scienza e medicina di base lavorino insieme per dare risposte concrete, alle famiglie e a tutti i pazienti, in modo particolare ai piccoli pazienti. un provvedimento che ha tenuto conto, giustamente, come si fa e come si deve fare sempre in questi casi, sia delle conoscenze scientifiche e accademiche su celiachia e diabete sia delle esperienze maturate da parte di chi vive sulla propria pelle pelle tutto questo, ovvero i pazienti e le loro famiglie. Prendiamo atto con soddisfazione che su questi temi c'è stata un'attenzione trasversale dei partiti e delle istituzioni. Vorrei ringraziare di cuore, per il grande e proficuo lavoro svolto, il ministro della salute Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato, la Commissione sanità, il presidente Zaffini e quindi tutto il Governo, per la sollecitudine con cui hanno seguito questo provvedimento, assicurando, dato non trascurabile, come abbiamo appena evidenziato, le prime necessarie e fondamentali coperture finanziarie, senza le quali una legge rischia di rimanere lettera morta. Ci sono battaglie che non hanno colori politici. La battaglia per la tutela della salute dei nostri cittadini, soprattutto dei pazienti affetti da celiachia e diabete di tipo 1 in età pediatrica, è certamente una di queste. Quando si tratta del bene degli italiani e della salvaguardia del principio della tutela della salute non possiamo e non dobbiamo dividerci, e abbiamo appunto visto i voti unanimi di quest'Assemblea. Ecco perché il voto di oggi assume un significato speciale: è una vittoria che appartiene a tutti, a partire dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie. L'Italia si appresta a tagliare un importante traguardo normativo e si pone all'avanguardia nella prevenzione di queste due patologie. In conclusione, quella che approviamo oggi è una buona legge, giusta, concreta e condivisa.

Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare oggi riguarda la prevenzione, destinata soprattutto alla popolazione di età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti a rischio di sviluppo di diabete di tipo 1 e di celiachia. La diagnosi precoce di queste due patologie che spesso aggrediscono i più piccoli è necessaria e dev'essere sostenuta per ridurre le complicazioni, potenzialmente mortali, che ne possono derivare. È importante intervenire in anticipo intervenire in anticipo e prevenire gli effetti dannosi sull'organismo di tipo irreversibile, tanto più che spesso i sintomi sono lievi, almeno in un primo momento. La correlazione tra le due patologie è molto studiata ed è importante che siano coinvolte le associazioni dei familiari e le fondazioni maggiormente rappresentative delle persone che ne soffrono. Diabete e celiachia e celiachia hanno in comune il fatto di essere due patologie che condizionano l'alimentazione - vorrei sottolineare questo punto - e condividono una similitudine anche nella gestione. Ci sono regole restrittive che devono essere seguite pedissequamente per mantenere un buon stato di salute, è fondamentale aderire a una dieta equilibrata e la distribuzione dei nutrienti dev'essere rispettata ad ogni pasto. Ne approfitto per portare all'attenzione dell'Assemblea un dato che impone una riflessione. L'Italia si colloca al secondo posto in Europa per diffusione dell'obesità infantile tra i maschi (21

non riescono ad alimentarsi in modo adeguato, dato che, come dicevano prima, queste patologie richiedono un certo tipo di alimentazione. Questa situazione di certo non migliorerà nei prossimi mesi, visto che a molte famiglie che vivono nella totale fragilità e nella povertà è stato addirittura tagliato il reddito di cittadinanza. Domando quindi: come potranno queste famiglie provvedere

possono segnalare l'insorgenza del diabete di tipo 1 o della celiachia. Durante i lavori in Commissione abbiamo avuto la possibilità di ascoltare i medici e i tecnici che hanno sviluppato tecnologie e strumenti diagnostici

tra l'altro con uno *screening* su base nazionale, costituisce un grande strumento di aiuto anche per chi poi queste patologie le deve vivere e per i nuclei familiari delle persone che ne sono affette, perché spesso si scoprono in maniera del tutto casuale o vengono all'evidenza con un fatto drammatico, come spesso succede ai bambini ai quali viene diagnosticato il diabete di tipo 1: vanno incontro a una crisi glicemica, poi a un ricovero e da lì a un'infausta diagnosi. Uno *screening* precoce consente anche alle famiglie di capire il tipo di vita che si dovrà fare e la terapia che si dovrà intraprendere e di accompagnare il bambino in questo percorso di vita, che è molto condizionante condizionante per le terapie che vanno fatte, per il tipo di attività e per l'adattamento metabolico che il soggetto deve fare prima di trovare una sua stabilità con la terapia insulinica, con tutto quello che ne consegue e che riguarderà il prosieguo di tutta la sua esistenza.

ma serve a sviluppare gli ulteriori strumenti che ci consentiranno - e questo è l'augurio che ovviamente tutti noi ci facciamo - di sconfiggere queste malattie, prevenendole davvero ed evitando che insorgano. I dati sono veramente drammatici, rilevando che sono circa 530.000 le stime di casi diagnostici di celiachia e di diabete di tipo 1. Probabilmente però il numero di persone effettivamente affette da questa patologia è anche superiore, perché molti fino a quando non si verifica l'evento scatenante, che avviene in modo casuale, non lo sanno e convivono con una patologia che silenziosamente comunque corrode il loro organismo fino a quando non si disvela in maniera drammatica. maniera drammatica. Accanto a questo *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica che è fondamentale e che incontra assolutamente il nostro pieno apprezzamento e sostegno, altrettanto importante è che si lavori per una opportuna promozione degli stili di vita, dell'educazione alimentare e del contrasto all'obesità, favorendo ancor di più, come già abbiamo fatto in Parlamento, l'attività sportiva. Allo sport abbiamo attribuito infatti il valore e il rango di principio costituzionale, proprio perché in esso individuiamo i valori sani sani del vivere civile, della capacità di sviluppare le inclinazioni naturali e di correggere abitudini sbagliate, favorendo una vita più sana.

sulla ricerca. Crediamo fortemente nella ricerca e la incoraggiamo sempre di più, perché, se vogliamo davvero migliorare la vita delle persone, bisogna puntare sugli strumenti di prevenzione e di contrasto. Accanto poi alla prevenzione e alla ricerca, c'è da valorizzare sempre di più la medicina di prossimità, affinché l'équipe medica non lasci mai sole le persone affette da patologie e soprattutto sostenga anche le famiglie nell'affrontare gli esiti e le conseguenze di tali

è un fatto importante. Quando parliamo di malattia, di salute e sanità, non avere barriere ideologiche è molto importante e continuare nel solco della prevenzione è sicuramente fondamentale. Il diabete, come sappiamo, è una delle malattie croniche più frequenti nell'infanzia e nell'adolescenza. Sappiamo altresì che dopo il Covid la celiachia purtroppo ha sviluppato numeri molto alti in età pediatrica e non solo. In modo particolare in Italia, la forma più diffusa di diabete in età evolutiva è rappresentata proprio dal diabete di tipo 1, pari a circa il 90 Nel mondo ci sono circa 1,2 milioni di bambini e adolescenti che hanno il diabete di tipo 1 e la maggior parte proprio nell'età sotto i quindici Il diabete di tipo 2, che fino a qualche anno fa rappresentava circa l'uno per cento dei casi di diabete in età pediatrica, è in progressivo aumento, come ci dicono anche gli ultimi dati di cui disponiamo. disponiamo. Sono numeri che pesano sul sistema sanitario e sociale e hanno un impatto molto forte non solo sul paziente, ma sulle famiglie. Nel 1997, come sappiamo, è stato istituito il Registro italiano di diabete insulinodipendente, proprio con lo scopo di raccogliere i dati epidemiologici sui nuovi casi di diabete di tipo 1. tipo 1. Bisogna continuare con tutti gli strumenti che abbiamo e rafforzarli affinché la prevenzione sia lo strumento su cui il Parlamento e il Governo continuino a legiferare e a monitorare. Tutto questo evidenzia comunque la necessità di un'attenzione istituzionale che, ancora di più in questo momento, deve avere grande importanza. Per fare questo, ovviamente, serve un approccio multidisciplinare, perché sappiamo che necessita di competenze e di specializzazioni importanti da quanto sappiamo, bisogna anche rafforzare e insistere sui centri di diabetologia pediatrica, perché questo poi significa avere un percorso di assistenza per aiutare ad avere soprattutto adulti sani, con ricadute positive sul sistema sanitario e sociale.

ma se pensiamo che malattie come queste hanno bisogno di un intervento prima di tutto preventivo, dobbiamo lavorare su questo. Sicuramente c'è da rivedere molto anche nella riforma sociosanitaria - a me piace chiamarla così ma dobbiamo farlo. Le Regioni sono al collasso e c'è la necessità di investire risorse nel sistema sanitario. Non si tratta soltanto difendere il diritto alla salute e i livelli essenziali di assistenza, che oggi non sono uguali in tutta Italia, anzi, dopo il Covid sappiamo che molte aree geografiche hanno differenze enormi, quindi ci sono un *deficit* e la necessità di investire sul personale medico e infermieristico, sugli operatori sociosanitari, sui consultori, sulle malattie e sulle nuove malattie rare. C'è da mettere a sistema un problema che ci portiamo avanti da troppi anni, che evidentemente non appartiene solo a questo Governo. Nella legge di bilancio dobbiamo fare questo sforzo: non è possibile

parlando ai bambini e alle fasce cosiddette più deboli e fragili e potremmo fare davvero quel salto di qualità che oggi serve al sistema sanitario in generale. Non è

Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese bellissimo anche dal punto di vista climatico, pertanto dobbiamo investire molto sul benessere della persona: si vive di più, ma si deve vivere meglio. Abbiamo la necessità di un percorso assistenziale che possa accompagnare il soggetto da quando nasce fino all'età adulta e poi nella fase di invecchiamento. Solo in questo modo potremo potremo parlare di un bene comune e di una difesa della comunità dal punto di vista sanitario, ambientale e sociale. Abbiamo tanti strumenti Spero che il Ministro abbia già espresso parere favorevole anche ad una nostra proposta di legge che riguarda il riconoscimento dello sport come farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica, su cui stiamo lavorando già dalla scorsa legislatura: è un altro tassello che può aiutare in questa riforma sociosanitaria che auspichiamo. Occorre garantire l'accesso alle possibilità di cura più appropriate, innovative e meno invasive, perché questo è un altro aspetto che ci interessa garantire ambienti ospedalieri e ambulatoriali accoglienti, adatti all'infanzia e all'adolescenza; assicurare sempre un gruppo multidisciplinare all'interno dei centri specializzati, dove medico di base, pediatra e altre figure fondamentali possano lavorare assieme; favorire un'azione di rete sul territorio tra centri di diabetologia pediatrica di riferimento regionale, centri di diabetologia dell'adulto, centri periferici, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale; facilitare la transizione della persona con diabete in età evolutiva dal diabetologo pediatrico al diabetologo dell'adulto. Abbiamo quindi la necessità di investire ancora di più nella scelta, con obiettivi chiari e scelte terapeutiche. L'ultima L'ultima è aiutare le famiglie in questo percorso di assistenza, sia per i bambini e gli adolescenti che hanno il diabete di tipo 1 (ma non solo), sia quelli affetti da celiachia. Dobbiamo fare un investimento su quest'ultima malattia, che è in continuo aumento, affinché anche le cure e i farmaci siano a buon mercato, perché oggi anche da questo punto di vista ci sono diseguaglianze sociali ed economiche che fanno la differenza.

alle cure preventive: questo sappiamo cosa vorrà dire in futuro, ma lo stiamo già vivendo nel presente. *(Applausi)*. Per tutte queste ragioni, mi appello ancora una volta al Governo.

Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, innanzitutto ci tengo a ricordare che il disegno di legge che è giunto all'esame dell'Assemblea è stato presentato dal deputato di Forza Italia, nonché vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, sin dall'inizio della diciannovesima legislatura. Non si tratta qui di rivendicare la primogenitura del disegno di legge, bensì

Camera. Vanno qui resi i dovuti ringraziamenti anche al ministro Schillaci, per la sua consueta disponibilità e competenza e per il fatto di aver reso concrete e attuabili le misure, mettendo a disposizione anche tutte le opportune risorse finanziarie, che in un disegno di legge come questo sono molto importanti.

Le modifiche introdotte alla Camera prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni e l'ascolto delle associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e celiachia. Il ruolo delle associazioni è fondamentale; è uno strumento straordinario, perché sprona il Parlamento, quindi tutti noi, ad approvare norme concrete concrete basate sulla loro esperienza, perché ovviamente, lavorando negli ospedali, sono a contatto direttamente con le patologie e quindi mettono in atto delle soluzioni ai problemi di salute. esame prevede che sia adottato un programma di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, a partire dal 2024. Viene inoltre istituito un osservatorio nazionale, composto da 13 membri che abbiano comprovata esperienza su questi temi. Si affida quindi alla scienza e alla ricerca un compito importantissimo, quello di studiare ed elaborare le risultanze dello *screening*, al fine di arrivare a una riduzione e al controllo degli effetti delle due patologie anni (come dicevo poc'anzi). Allo stesso tempo, si avvia una campagna di sensibilizzazione sociale, anch'essa realizzabile concretamente in quanto dotata delle opportune autorizzazioni di spesa e coperture finanziarie. Se me lo consente, Presidente, vorrei rileggere le parole del presidente Mulè, che ha spiegato alla Camera la ragione di questo disegno di legge e - aggiungo io - la necessità di approvarlo al più presto: questa legge nasce grazie alla storia di due ragazzi: uno si chiamava Alessandro, l'altro si chiama Alfonso. Hanno la stessa età, hanno tredici anni, entrambi studenti di terza media, la stessa città di residenza, la stessa patologia (il diabete di tipo 1), ma un destino diverso. Alessandro non è più tra noi perché non gli venne diagnosticata in tempo una forma acuta e grave di chetoacidosi diabetica, che è la più comune tra le complicanze legate al diabete di tipo 1.

Nonostante fosse sottoposto allo *stress* degli esami di terza media, aveva le gambe che gli pesavano come se fossero dei macigni, come se qualcuno lo avesse bastonato e aveva una sete inarrestabile, continua. La fortuna di Alfonso - se così la possiamo chiamare fu che, fin dall'età di due anni, sapeva di essere celiaco e, dunque, quei sintomi furono ricollegati a una degenerazione della patologia con insorgenza di diabete di tipo 1 attraverso quella crisi di chetoacidosi. Alfonso si è salvato e oggi convive con la patologia grazie alla straordinaria capacità che lui ha (come ce l'hanno decine di migliaia di ragazzi) di saper convivere con una vita che è stravolta. Nessuno lo potrà mai sapere, ma se questa legge fosse stata già in vigore alcuni anni fa, c'è la ragionevole certezza che Alessandro non sarebbe morto. sarebbe morto. Cosa voglio dire? Con gli *screening* che verranno realizzati riusciremo a salvare altre vite di incolpevoli ragazzini, posto che quattro ragazzi ogni giorno scoprono di avere il diabete di tipo 1, mentre un ragazzo ogni 60 scopre di essere affetto da celiachia. Il testo oggi in esame in Aula non verrà modificato e consentirà alle norme che sono in esso contenute di entrare in vigore il più presto possibile, salvando così altre vite.

Non è la prima volta che capita quando si tratta di sanità, forse è la prima volta in questa legislatura (non ho tenuto il conto), ma di certo è capitato diverse volte nella

quando in realtà alla sanità ne servirebbero 10 o 15 e sarebbe stato bello se anche per questo ci fossimo messi a lavorare tutti insieme intorno a un tavolo per trovare quelle risorse così necessarie, perché quattro miliardi sono davvero il minimo per non sprofondare e non mandare il nostro sistema sanitario a gambe all'aria. Mi sembra quindi fondamentale che si trovino, ma sarebbe bello trovarne di più, perché il definanziamento del nostro sistema sanitario è qualcosa a cui speravamo di non assistere più

dovrebbe essere un pilastro fondamentale della nostra sanità, perché tutti noi sappiamo che ogni euro speso in prevenzione è un investimento sul futuro, non solo della salute degli individui, ma sul futuro del nostro perché le risorse che spendiamo in prevenzione sono soldi risparmiati su *welfare,* sulla previdenza sociale, soldi che l'INPS non dovrà erogare per pensioni di invalidità o altro tipo di assistenza nei confronti di cittadini che hanno dei problemi e che quindi non possono lavorare del tutto o abbastanza per mantenersi in maniera dignitosa; sono soldi che pesano sul sistema famiglia, perché ogni persona non autosufficiente ha accanto a sé (quando è fortunato) un *caregiver* che si prenderà cura di lui e che quindi comunque non potrà svolgere pienamente un'attività lavorativa. sappiamo che sono un impegno per il futuro del Paese, ma ancora non riusciamo a cambiare il paradigma

non sono spesa corrente ma, appunto, investimenti. Mi auguro che tutti insieme, così come stiamo andando verso l'approvazione di questo fondamentale disegno di legge per la vita di tantissimi tantissimi bambini di oggi che saranno cittadini di domani, riusciremo anche a portare a meta un altro importante lavoro sulla diversa classificazione di queste spese. Non mi dilungo sui dettagli del provvedimento in esame, perché già ne hanno parlato benissimo le colleghe che mi hanno preceduto. L'impegno per la tutela della salute dei nostri bambini dovrebbe essere il primo obiettivo: in questo caso lo raggiungiamo e possiamo spuntare questa casella. Spero che i prossimi provvedimenti che potremo esaminare insieme abbiano un respiro più generale e trasversale, invece di intervenire sempre con interventi con interventi normativi puntiformi, che però lasciano inalterato un sistema che comincia a fare acqua da più parti. Invece tutti insieme dovremmo capire che la prevenzione non riguarda solo questi aspetti, che il potenziamento delle strutture territoriali vale per queste come per tutte le altre patologie e per tutti gli altri cittadini che ne hanno bisogno e che, per esempio, la transizione dall'età pediatrica all'età adulta dei nostri bambini con patologie croniche riguarda sicuramente i bambini affetti da diabete di tipo 1 o da celiachia, ma non solo loro. Lo stesso discorso lo potremmo fare infatti per i bambini che sono stati sottoposti a un trapianto, così come per tantissime altre patologie. Quindi mi auguro che in futuro riusciremo ad avere una visione sul sistema salute più trasversale e strutturale, che ponga finalmente rimedio ad alcuni problemi che ci trasciniamo da anni e che restano ancora irrisolti. Nonostante questo, per le ragioni che ho già esposto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La proposta di legge in votazione prevede infatti di spingere il processo di prevenzione nella popolazione pediatrica, da uno a diciassette anni, del diabete di tipo 1, con lo scopo di evitare complicanze lesive sulla salute dei pazienti. Il provvedimento, attraverso un attento *screening* predittivo, consentirà una maggiore informazione sulle cause di insorgenza della malattia e l'inserimento precoce di terapie farmacologiche che ne rallentano il corso. Altrettanta Altrettanta attenzione viene data alla diagnosi precoce della celiachia, causa di complicanze gravi, se non diagnosticata. Le due patologie in oggetto non a caso sono state accoppiate, perché hanno dei profili di omogeneità, nella eziologia, nell'insorgenza e nella platea di riferimento. Il diabete di tipo 1 rappresenta circa il 10 per cento dei soggetti diabetici ed è chiamato spesso diabete giovanile o insulino-dipendente, in quanto insorge proprio nell'infanzia e nell'adolescenza. È una malattia cronica più frequente nell'età pediatrica, si stima circa attorno all'85-90 da diabete di tipo 1 sono circa 300.000. Invece, per quanto riguarda la celiachia, è stato calcolato che nella popolazione il numero totale dei celiaci sia di circa 600.000, ma ne sono stati diagnosticati solo 241.729. Questi sono gli ultimi dati, secondo la relazione

Ecco perché diventa importante sempre più diagnosticare questi casi, che sono in crescita. I dati relativi al 2022 parlano di 10.210 nuove diagnosi, con una prevalenza della Bisogna considerare anche la quantità e la qualità importante di complicanze che potrebbero generarsi a causa della mancata diagnosi: penso al diabete, alla chetoacidosi, alle malattie cardiovascolari, alle neuropatie, alle neoplasie, alle complicanze oculari, alle amputazioni. Per i celiaci in età pediatrica, ciò potrebbe comportare una flessione del ritmo accrescitivo, un ritardo della pubertà e dello sviluppo e un malassorbimento intestinale in età giovanile, fino ad arrivare direttamente a malattie importanti quali il tumore o a conseguenze appunto

diagnosi, quindi, perché è una patologia cronica, evolutiva e ad alto rischio di complicanze: chi ne è affetto avverte tutto il disagio per le conseguenze che ne derivano e c'è il timore di una vera e propria rivoluzione nella quotidianità. Per questo si parla di malattie sociali: provate per un giorno o solo per un pasto a fingere di essere celiaco e a entrare in un bar, in un ristorante, in un ambiente pubblico o a viaggiare e provate a chiedere un pasto oppure uno spuntino senza glutine e vedrete la risposta oppure l'ampia scelta - per modo di dire - che vi viene sottoposta.

che ringrazio, per andare a modificare la legge n. 123 del 2005 sulla celiachia, per implementare la dematerializzazione e la circolarità dei buoni per i prodotti senza glutine, affinché si possa uniformare la loro erogazione su tutto il territorio italiano, grazie a un investimento programmato con i fondi del PNRR volto a potenziare il fascicolo sanitario elettronico e il sistema della tessera sanitaria. L'altro impegno assunto riguarda il sostegno alla formazione della classe medica, come dicevo, delle professioni sanitarie e degli operatori del settore Horeca e naturalmente anche alla formazione nelle scuole alberghiere proprio per fare informazione. Tornando al disegno di legge in discussione, si istituisce anche un osservatorio sul diabete di tipo 1, con il compito di elaborare le risultanze sullo *screening* e favorire campagne importantissime di sensibilizzazione e di formazione. Lo *screening*, combinato con la stessa indagine, individuerà in via predittiva i soggetti a rischio patologico di celiachia e diabete di tipo 1. La prevenzione è sicuramente un tema di politica sanitaria attuale e moderna, sia in termini di adeguatezza delle cure che di risparmio di risorse e si inserisce in un contesto di razionalizzazione delle risorse economiche, ma ancora di più di promozione del sistema sanitario nazionale in termini di tutela della salute, specialmente in età pediatrica Lo *screening* del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca, quindi, l'istituzione di questo osservatorio, le campagne di sensibilizzazione e di formazione mostrano l'attenzione del Governo ai temi di salute e di sanità pubblica ed è per questo che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito

che questo provvedimento si debba approvare. È raro che la politica sia capace di trovare una certa trasversalità, ma quando si discute di temi che hanno a che fare con la vita delle persone, lo si deve provare a fare sempre in esame è un provvedimento che con la vita delle persone ha una certa attinenza. Grazie all'approvazione di questa legge, infatti, prevediamo e finanziamo la possibilità di effettuare diagnosi precoci in casi nei quali altrimenti il pericolo e le conseguenze sarebbero potenzialmente mortali. Ecco perché il legame con la vita, perché in questo modo agiamo prima, preveniamo nel migliore dei casi, la salviamo. Come è stato detto, in Italia ogni giorno quattro bambini scoprono di essere affetti da diabete di tipo 1, una patologia che in molti casi ha carattere asintomatico e che quindi viene scoperta quando ha già fatto dei danni. Con lo *screening* arriviamo prima, individuando precocemente la malattia, il che ci permette di prevenire e, dunque, non solo di curare meglio, ma anche di sgravare il nostro sistema sanitario nazionale dai costi legati a un intervento successivo, tardivo e, appunto, più costoso. Anche sulla celiachia, ovviamente, il passo avanti è evidente, perché questa legge ci consente di fotografare ed individuare un problema che troppo spesso non emerge, per una sintomatologia assente oppure estremamente lieve. Quando ci si accorge di essere celiaco molto spesso si è in una fase nella quale si è già messo sotto stress l'organismo, che nel frattempo lamenta disturbi gastrointestinali e spesso patologie ancor più gravi. più gravi. Come legislatori, possiamo dire di aver fatto un buon lavoro quando, grazie al nostro impegno e grazie ad una legge da noi approvata, la vita dei nostri concittadini migliora. penso che questo provvedimento cambierà la vita, non solo a migliaia di persone malate, ma anche a migliaia di famiglie e genitori che sono chiamati a gestire la vita di chi è affetto da una malattia come il diabete

Sappiamo tutti cosa significa, in una famiglia, dover rispettare le esigenze e i ritmi di chi ha una malattia come questa. Anche per questo, mi unisco ai ringraziamenti alla Fondazione italiana diabete, che so essere stata in prima linea per il conseguimento di questo risultato. Ringrazio i colleghi deputati, che questo provvedimento hanno presentato, discusso e approvato. A noi spetta il compito di renderlo un atto di legge e, come Partito Democratico, non faremo mancare il nostro sostegno affinché questo avvenga. Pur tentando di non rompere questo clima di idillio, ci terrei però a fare un appello al Governo e a tutta la maggioranza.

Come dicevo prima, questa legge salva la vita di migliaia di persone. Ebbene, signor Presidente, mi lasci dire che l'investimento nel sistema sanitario pubblico serve ad essere orgogliosi di avere gli strumenti per salvare la vita di milioni di persone, per migliorarla, per allungare sempre di più la speranza di vita di chi sta male. Per questo motivo siamo d'accordo con la richiesta avanzata dal ministro Schillaci, di dedicare al capitolo sanitario ulteriori quattro miliardi di euro rispetto a quelli previsti dal Documento Siamo convinti che non bastino, ma sarebbe già un buon inizio. Il Governo si assuma l'impegno di farlo subito, in maniera molto più consistente e, se possibile, nella stessa legge di bilancio. Se farete questo ci troverete con lo stesso atteggiamento che abbiamo tenuto oggi: positivo e collaborativo. Lo facciamo anche forti del fatto che, quando eravamo al Governo e Ministro della salute era Roberto Speranza, il Fondo sanitario nazionale è stato finanziato al 7 per nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Avevamo tutti detto, anche chi allora era all'opposizione, che avevamo imparato la lezione, che il Servizio sanitario nazionale non sarebbe stato mai più sotto finanziato, ma non è quello che risulta nel DEF. Noi abbiamo assoluto bisogno che i cittadini italiani e gli operatori socio sanitari ricomincino a credere nel nostro Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo evitare la fuga generale dei medici dal Servizio sanitario nazionale e riaprire una discussione definitiva che porti all'eliminazione dei tetti alla spesa del personale nella sanità, anche con l'obiettivo di pagare di più i nostri operatori. Siamo anche pronti a sostenere qualsiasi azione per l'attuazione della missione 6 del PNRR. Su questo, devo confessare che sono particolarmente preoccupata, perché l'ultimo documento del Governo su questa materia presenta tagli al finanziamento per la realizzazione di ospedali e case di comunità: peraltro senza nemmeno dire quali e probabilmente arrivando a tagliare strutture la cui costruzione è addirittura già partita. Non dite che mancherebbe il personale per far funzionare queste strutture, perché il ministro Speranza aveva ottenuto che il personale da assumere per la medicina territoriale sarebbe stato al di fuori del tetto di spesa: ve lo voglio ricordare. perdonare nessun ritardo, perché nessun ritardo sarebbe giustificato e giustificabile quando si parla della cura e della presa in carico dei nostri concittadini. Togliere dal pronto soccorso pazienti che possono essere curati altrove consente di alleggerire la situazione e ai medici di concentrarsi meglio sui pazienti che hanno più bisogno. Proprio per questo l'Europa ci ha dato i soldi. Nemmeno sarebbe Nemmeno sarebbe accettabile un altro modello di sanità diverso da quello che abbiamo conosciuto finora - ovviamente mi riferisco al servizio sanitario pubblico e universalistico - perché sono sicura che nessuno di voi, colleghi della maggioranza, approvi il modello che chi che chi può pagare salta la fila al pronto soccorso. Durante questo dibattito si è parlato di prevenzione, di *screening*, di possibilità di tenere traccia delle condizioni di salute dei malati. Ecco, la pandemia su questo ha segnato un punto dal quale dovremmo trarre insegnamento o almeno avremmo dovuto: dove si è investito su una sanità pubblica, capillare, strutturata, connaturata con i servizi socioassistenziali, la risposta del tracciamento e la stessa capacità di prevenzione sono state decisive. Allora, vi prego, non torniamo indietro: è un appello sincero che però temo cadrà nel vuoto, e mi sembra davvero assurdo. tornando sul provvedimento che ci accingiamo a votare, per segnalare un altro aspetto che trovo importante: è una legge di iniziativa parlamentare che arriva al traguardo - ahimè - in solitaria, ma è la dimostrazione che, se c'è la volontà politica, il Parlamento può tornare a svolgere le funzioni costituzionalmente previste e garantite. Di provvedimenti di questa natura ce ne sono diversi e su tutti sarebbe bello avviare una discussione seria, senza relegare queste Aule al mero lavoro di conversione dei decreti-legge d'urgenza. Nel frattempo, con il voto favorevole di tutto il Gruppo Partito Democratico siamo convinti di dar forza e sostanza a questo provvedimento. *(Applausi)*.

È proprio con la prevenzione che si attua una politica sanitaria moderna, sia in termini di adeguatezza delle terapie che di risparmio di risorse; tutto ciò è ancora più vero quando si tratta di patologie dell'età pediatrica. Quello in esame è infatti un programma di *screening* predittivo di ricerca ematologica di autoanticorpi specifici che deve agevolare la diagnosi precoce, e di conseguenza ridurre l'incidenza delle potenziali complicanze, del diabete di tipo 1 e della celiachia in età pediatrica, in particolare nella fascia di età che va da uno a diciassette anni. Come già ampiamente ricordato, il diabete tipo 1, il diabete giovanile, è una patologia cronica endocrino-metabolica che rappresenta circa il 10 per cento delle forme di diabete ed è molto più frequente nell'età pediatrica, dove rappresenta oltre l'80 dei casi di diabete in età evolutiva, mentre la celiachia è un'enteropatia autoinfiammatoria permanente, con tratti di autoimmunità, scatenata dell'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di patologie dai numeri rilevanti: infatti si stimano in 300.000 i casi diagnosticati di diabete di tipo 1 e in circa 230.000 i casi di celiachia, con circa 11.000 nuove diagnosi annuali. Inoltre, l'incidenza del diabete di tipo 1 è purtroppo in progressivo aumento in tutto il mondo e in Italia, dove ne è affetto circa lo 0,5 per cento della popolazione, ha una prevalenza che è raddoppiata negli ultimi venticinque anni ed è in ulteriore e costante incremento.

Ci troviamo quindi davanti a patologie non sempre correttamente riconosciute precocemente, spesso anche a causa di una sintomatologia iniziale di lieve entità o atipica, con la conseguente mancanza di un'adeguata e tempestiva appropriatezza terapeutica e del rischio di insorgenza di complicanze, a volte anche molto gravi, quali per il diabete la chetoacidosi, già ricordata ampiamente, complicanze cardiovascolari, la neuropatia diabetica, la nefropatia diabetica e le complicanze oculari come la retinopatia diabetica.

Entrambe le patologie quindi possono evolversi con complicanze gravi ed invalidanti che possono essere ridotte notevolmente con una diagnosi precoce e una corretta terapia e che, viceversa, possono essere aggravate e accelerate dalla non aderenza alla terapia insulinica per i diabetici e da una non corretta dieta priva di glutine per i celiaci. Va inoltre sottolineata la validità della scelta di accoppiare le due patologie in questo provvedimento. Infatti esse presentano dei profili di omogeneità sia nell'eziopatogenesi autoimmunitaria sia nell'età di insorgenza ed esiste un'ampia e consolidata letteratura che mette in evidenza una possibile correlazione fra le due forme morbose con una prevalenza di associazione che va dal 4,1 al 6,5 per cento. È pertanto corretta la scelta di un doppio *screening* diabete-celiachia per le evidenze scientifiche di una possibile comorbilità. Venendo all'articolato, esso prevede all'articolo 1 un termine di centoventi giorni per l'emanazione di un decreto del Ministro della salute che detti criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale da avviare a decorrere dall'anno 2024 per l'individuazione degli anticorpi del diabete tipo 1 e della celiachia, finalizzato a prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete tipo 1. 1. Al comma 2 si autorizza l'attuazione di un programma pluriennale la cui spesa è pari a 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. All'articolo 2 è prevista l'istituzione presso il Ministero della salute di un osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, composto da 13 membri da nominare con decreto del Ministro della salute, dove sono presenti anche due rappresentanti per ciascuna patologia delle associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari. È questa una presenza importante per i risvolti sociali e psicologici che investono le famiglie dove è presente una persona affetta da queste patologie croniche. Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale ad opera del Ministero della salute, promuovendo campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza dei programmi di *screening*. In conclusione questo provvedimento, colleghi, rappresenta certamente un esempio che pone al centro delle politiche sanitarie la prevenzione, un tema che in questi mesi è stato sempre una priorità dell'attività di Governo con diverse iniziative promosse dal Ministero della salute. La prevenzione deve essere sempre considerata un investimento con un ritorno in termini di sostenibilità e di risparmio per il sistema del Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto un investimento per i pazienti e le loro famiglie. Desidero concludere affermando come un voto favorevole ampiamente condiviso su questo provvedimento, così come è avvenuto presso la Camera dei deputati, sia un importante segnale di attenzione e vicinanza a quanti, pazienti e famiglie, vivono quotidianamente il dramma della situazione della malattia cronica. Annuncio pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

viene decantato soprattutto per la presa in carico dei costi - perché avere celiachia e comporta anche spesso l'impoverimento della famiglia - e perché vi si parla di terapie fisiche precoci. Mi permetto di aggiungere che la cosa più importante di tutte è la presa in carico psicologica, perché queste patologie tendono a ferire il corpo, ma soprattutto a ferire la psiche dei bambini, degli adolescenti e degli adulti per i quali una presa in carico psicologica, seria e professionalmente

parlare di benessere e non solo di assenza di malattia, che credo sia importante. Viva il corpo, ma soprattutto viva l'anima, in un dualismo perfetto.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022,

dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023. Inoltre il provvedimento, composto da 14 articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità, del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono infine conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica». Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato, n. 833, non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito

alle tante ricordate, anche ieri, dal Presidente della Repubblica, associandoci alle sue parole sulla necessità che tutti, Governo, maggioranza, opposizione e qualunque organismo dello Stato, facciano di più per contrastare questo stillicidio di morti, di tragedie, che colpisce fortemente non solo la nostra umanità, ma la convivenza civile della nostra Nazione. Su questo tema, credo che tutti sentiamo la necessità di unirci e di sottolineare l'obbligo di fare sempre di più, tutto quello che si può fare. In ricordo delle nuove tre vittime e degli altri caduti negli incidenti di lavoro, vi prego di voler condividere insieme un momento di cordoglio, rimanendo per qualche secondo in silenzio.

Signor Presidente, ringrazio il Governo e i Ministri presenti, tutti i senatori e le senatrici.

ha deciso di dedicare una seduta di discussione al tema della sicurezza. Oggi, purtroppo, siamo di fronte a un'altra tragedia, ma vorrei ricordare che la media è di tre morti al giorno. Sostanzialmente, siamo in questa situazione.

per l'impostazione di un programma di lavoro che la Commissione doveva porsi, e si deve porre. Di fronte alla tragedia di

unitaria di discussione e risoluzione. Abbiamo cercato di lavorare in questa direzione e qui voglio davvero ringraziare tutti i membri della mia Commissione, perché tutti hanno dato un contributo e insieme

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le morti bianche rappresentano una piaga nella nostra Nazione: ogni vita persa sul luogo di lavoro non solo ha un impatto devastante sulle famiglie coinvolte, ma influisce anche sulla società nel suo complesso. Ogni incidente mortale rappresenta un costo sociale ed economico in termini di assistenza sanitaria, indennizzi, disabilità permanente e perdita di produttività. I dati forniti dall'INAIL - lo ricordava prima il senatore Tino Magni - da gennaio a luglio riscontrano un bilancio ancora fortemente drammatico: 559 vittime, con una media di 80 decessi al mese e un aumento del 4,4 per cento in più rispetto all'anno scorso. Ma si tratta di vite umane perse, famiglie distrutte e comunità che soffrono. È dunque una questione che richiede la nostra totale attenzione e delle azioni concrete. Il problema al quale oggi cerchiamo di dare risposta è pertanto di estrema importanza e rappresenta, prima di tutto, una battaglia di civiltà. La sicurezza dei lavoratori è un tema già al centro dell'agenda di Governo, che ha già mosso i primi passi in questa direzione, ad esempio incrementando per l'anno 2023 di 5 milioni di euro il fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ed estendendo la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, includendo anche quello della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambiti scolastici. Inoltre, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di formazione, come la nomina del medico competente e poteri di vigilanza volti a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste sono certamente scelte importanti di riforma normativa. Avremo modo di vederne i risultati sul medio e lungo termine, ma di fronte ai numeri che ho appena citato è sicuramente necessario implementare implementare ulteriori interventi, dal momento che ogni giorno migliaia di lavoratori si recano sul loro posto di lavoro con la certezza che la sera torneranno a casa dai loro affetti e dalle loro famiglie. Ma questa certezza viene distrutta con una media di tre volte al giorno da incidenti che spesso e volentieri si sarebbero potuti evitare. Come? Applicando protocolli di sicurezza corretti e semplici regole di buonsenso. Quando leggiamo alcune agenzie stampa - è di ieri sera quella di un operaio caduto da un ponteggio in un cantiere edile privato a Messina ed è di poche ore fa fa quella che citava il presidente La Russa, di due morti accertati nell'esplosione dentro una fabbrica abruzzese già interessata, fra l'altro, in passato da altri gravi incidenti - sembra che in settant'anni nulla abbiamo imparato da Marcinelle, ad esempio, dove i nostri operai furono di fatto condannati a morire in una miniera costruita come una trappola per topi senza vie di fuga, senza alcuna strategia per prevenire eventuali incidenti e alcun programma per provvedere ai soccorsi. Nel corso di questi decenni molteplici sono state le sentenze che hanno scoperchiato un mondo imprenditoriale dove gli operai vengono sfruttati fino a lavorare anche dodici ore al giorno e dove i sistemi di sicurezza non funzionano. Per alcune aziende la sicurezza è semplicemente un costo in più da cancellare in bilancio, una perdita di tempo, una trafila burocratica alla quale sottrarsi con furbizia. Dall'altro lato, alcune volte sono gli stessi operai a trascurare alcune norme di buonsenso. Si tratta, quindi, non solo di ragionare solo di leggi e di regolamenti, ma anche di promuovere una cultura della sicurezza. Si tratta di una presa di coscienza del valore della persona e di come proteggerla. Si tratta di promuoverla in ogni ambiente lavorativo. Si tratta del fatto che la tutela della vita diventi una priorità e che questa priorità sia condivisa da tutti. Pertanto, se è vero che noi, cari colleghi, abbiamo il dovere di registrare normative solide e rigorose che prevedano controlli severi e sanzioni efficaci per chi non rispetta le leggi, dall'altro dobbiamo anche patrocinare la cultura della sicurezza, introducendola nella formazione scolastica e invitando a investire sulla formazione obbligatoria tutti i lavoratori a tutti i livelli, affinché siano consapevoli dei pericoli e delle procedure per evitarli. Nessun lavoratore deve mai mettere a repentaglio la propria vita per guadagnarsi da vivere. Per concludere, è imperativo riconoscere che il tema cruciale discusso oggi non può più essere trascurato. Abbiamo l'opportunità di governare il processo per portare ad un'inversione di questo tragico *trend* e sono sicura che questa causa possa incentivare tutti noi ad unire le forze presenti in quest'Aula per accogliere positivamente questa mozione, che rappresenta non solo una sintesi *bipartisan*, la più rappresentativa possibile, ma anche un impegno che prevede azioni concrete a Nel ringraziare per l'importantissimo lavoro fatto dai colleghi della Commissione, credo che su un testo che parla di implementazione di normative efficaci, di investimenti sulla formazione e di un grandissimo impegno nel creare una coscienza della sicurezza non si possa che esprimere un sonoro e unanime «sì», uniti dalla consapevolezza che siamo qui a tutelare il bene più alto, che è quello della vita umana.

il presidente La Russa, aprendo la sessione pomeridiana, ha ricordato il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla ministra Calderone in occasione del corso di formazione sui nuovi ispettori di lavoro, - come veniva detto prima - sul fatto che non stiamo facendo abbastanza. Quel «non stiamo facendo abbastanza» è rivolto a tutti, tanto alla maggioranza quanto all'opposizione. motivo la mozione unitaria che è stata siglata oggi, per la quale ringrazio il presidente della Commissione di inchiesta Tino Magni per il lavoro che ha voluto fare, deve servirci, ognuno per la propria parte, a fare qualcosa di più rispetto al passato. come me e come il mio Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, cerca di interpretare il ruolo dell'opposizione in maniera costruttiva, fare di più significa anche cercare di portare avanti un linguaggio di verità che vada forse oltre le analisi che sono state fatte fino a questo momento. C'è un'altra parola del messaggio del Presidente della Repubblica che dovrebbe farci molto riflettere, oltre al «dobbiamo fare di più»;

Se noi immaginiamo che i morti e gli infortuni sul lavoro debbano essere contabilizzati (prima ci veniva ricordato: un morto ogni otto ore, un infortunio ogni minuto), rischiamo di pensare che sia una situazione di numeri che non riusciamo ad abbassare, ma che in qualche modo è stabile. Temo invece che quel numero sia più alto dei dati ufficiali: non facciamoci fuorviare dalla stabilità del dato INAIL, le cui tabelle non offrono un quadro completo del dramma, perché l'Istituto riceve solo le segnalazioni dei decessi dei lavoratori assicurati. Questo significa che ci sono più morti e più infortuni sul lavoro che non vengono comunicati e questi dati li trovate negli osservatori ufficiali e non ufficiali, che ci dicono che già oggi in questo momento il numero dei morti, per esempio, è superiore al migliaio. Altrimenti, come si farebbe, per esempio, a valutare il tema dei decessi dei lavoratori autonomi o delle Forze dell'ordine o di altre forze che non fanno parte in questo momento dei dati ufficiali dell'INAIL? Infine, c'è un tema che secondo me bisogna affrontare con maggiore verità, che riguarda tanto i morti tanto gli infortuni sul lavoro. Se assumiamo l'idea che una persona abbia bisogno di avere più formazione nella sicurezza sui luoghi del lavoro, più formazione sulle scuole, più formazione nel mondo dell'istruzione, sicuramente stiamo dicendo una cosa vera, ma se andate a vedere l'età di chi subisce un infortunio sul lavoro, scoprirete che magari era stato assunto il giorno prima. Forse bisogna avere il coraggio di dire che in quel caso non si tratta di un infortunio sul lavoro dettato da inesperienza, ma di lavoro nero. molti dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro si chiamano lavoro irregolare e lavoro nero *(Applausi)*, perché, quando una persona viene assunta il giorno prima di un infortunio, molto spesso dietro quell'assunzione c'è una minaccia, c'è l'idea che possa continuare a lavorare senza danneggiare l'azienda, ma attraverso la regolarizzazione del contratto di lavoro. Allora sì alla formazione, sì alla prevenzione, sì all'istruzione; ma per prima cosa noi dobbiamo contrastare, tutti insieme, il lavoro nero e irregolare, che è una piaga sociale

il tema delle norme ha bisogno di un *check up*, ha bisogno di fare una revisione. Dal 2008 ad oggi il mondo del lavoro è completamente cambiato: cambiato: subisce trasformazioni molto forti, molto radicali e molto accelerate, anche attraverso il tema della transizione digitale, sul quale tornerò, però anche nel linguaggio che usiamo dobbiamo fare uno sforzo in più. Io, per esempio, non penso che sia utile utilizzare l'espressione "morti bianche", perché non c'è niente di bianco in un morto sul lavoro. *(Applausi)*. Penso che non ci sia più bisogno di usare la parola "infortuni" sul lavoro, perché non c'è niente che riguardi una questione di fortuna o sfortuna: si chiamano lesioni. *(Applausi)*. Io penso che non abbiamo bisogno di nuove norme o di norme più severe; penso che abbiamo bisogno di applicare le leggi che già abbiamo. Questo significa avere memoria. Il 12 dicembre 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli ispettori del lavoro sono scesi in piazza, per chiedere - il Ministro lo sa - un adeguamento dei loro piani contributivi e dei loro piani retributivi agli altri elementi dell'amministrazione statale. Quella vertenza è stata parzialmente risolta, anche grazie all'intervento del Governo, al quale riconosco che sta facendo passaggi importanti. Se però il tema è quello della parità tra chi si occupa di sicurezza del lavoro e gli altri amministratori, noi dobbiamo fare un salto in più,

Cerchiamo di capire quanto sono forti le trasformazioni del mondo del lavoro. Non vorrei che ci rassegnassimo all'idea ineluttabile che questi sono i numeri e che noi non riusciamo a incidere. Se le nostre analisi sono sbagliate, allora anche le nostre proposte per risolvere quei problemi rischiano di essere inefficaci. E allora forse, più che nuove sanzioni, più che nuove pene o più che nuovi reati, quello che serve è dare risorse, strutture e personale a chi si occupa di controllo sulla regolarità nel lavoro, perché non sia svuotare il mare con un cucchiaio.

un altro elemento, che invece vuol essere di speranza, che è contenuto nella mozione e che è stato affrontato da tutti anche all'interno dei lavori della Commissione. Noi abbiamo detto: smettiamola di pensare che la transizione digitale riguardi, per esempio, solo l'applicazione del digitale l'applicazione del digitale nei processi produttivi. Proviamo a pensare che la transizione digitale e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e della strumentazione digitale e tecnologica possano servire per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Io sono rimasto sconvolto da un elemento che vorrei fosse di riflessione per tutti: possiamo capacitarci che nel 2023 l'unica strumentazione digitale a gestire la segnaletica di un tratto in cui stava passando un treno sia un telefono? Mi guardo e rivolgo la domanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: ministro Salvini, è giusta l'idea di mettere in campo tanti cantieri che possono sbloccare delle opere; è giusto lavorare sulla velocità dei lavori, ma io credo - e spero che lei sia di questo convincimento - che andare veloci sia utile quando la prospettiva è quella di andare lontani. Quando si sburocratizzano alcuni passaggi della filiera degli appalti e dei subappalti, il rischio è infatti che lì si possano annidare mancate risorse nella prevenzione e nella

Questa mozione deve riuscire a livello unitario a portarci tutti a fare un passo avanti: è quello che ci chiedono non solo le vittime, ma anche i familiari delle vittime nei luoghi di lavoro. Bisogna cioè rifiutare l'idea che la persona umana, il lavoratore, possa essere degradato a scarto produttivo, a costo. Se noi riusciremo a fare quest'operazione culturale, probabilmente ci muoveremo nel solco di quello che ci dice il Presidente della Repubblica, cioè che non stiamo facendo abbastanza e abbiamo il dovere tutti quanti di fare qualcosa in più.

e doloroso parlare oggi in quest'Aula, perché l'incidente da cui prende spunto questa mozione è avvenuto nella mia Provincia, a pochi chilometri da casa mia, e ha fatto riaffiorare il dolore che provammo tutti nel 2007, quando ci fu l'incidente della ThyssenKrupp sempre nel mio territorio e altre vite di lavoratori furono spezzate durante l'orario di lavoro, mentre pensavano

È quindi difficile per me intervenire oggi, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sentire tutti noi la responsabilità di quei morti. Dopo il 2007,

e che però non è stato abbastanza. Si pensava di aver raggiunto un grande traguardo con quel decreto legislativo e di aver finalmente posto un freno all'emorragia di vite, ma non è bastato, anche perché la cultura della sicurezza è rimasta sulla carta, in quanto ancora oggi mancano addirittura alcuni dei decreti che dovevano seguire a quel provvedimento.

non resti una bella dichiarazione di intenti, ma che ne derivino provvedimenti legislativi che facciano sì che i lavoratori la sera tornino a casa. Ci sono molte cose che possiamo fare e abbiamo detto tante volte che avremmo potuto farle, ma forse è arrivato finalmente il momento di farle, anche perché non abbiamo ancora finito di chiudere il capitolo relativo a quello che è accaduto a Brandizzo a fine agosto e oggi, purtroppo, ci siamo ritrovati

(ILN), più personale, perché sono anni che la contrazione delle assunzioni ha fatto sì che non ci fosse un adeguato ricambio in tutto il comparto pubblico. diciamo che i lavoratori pubblici sono fannulloni e poi ci troviamo qui a dire che ne dobbiamo assumere di più: non sono fannulloni, ma spesso non vengono messi nelle condizioni di lavorare bene.

infatti essere in grado di guardarsi intorno e di capire dove possono essere le criticità. Vanno inoltre implementati i dialoghi tra le banche dati

ci riguarda ogni giorno, in ogni istante, anche quando saliamo in macchina, magari su un sedile posteriore e non ci mettiamo la cintura di sicurezza, perché pensiamo che sia solo un fastidio, o quando mettiamo in macchina i nostri figli e non li assicuriamo nel seggiolino. Magari pensiamo che siano tutte assurdità, anche se siamo tutti abbastanza informati su quanto questi presidi servano a salvare delle vite. Eppure, penso che a ciascuno di noi capiti ogni tanto di voltare lo sguardo sulla macchina che ci sta accanto e di vedere magari un bambino di tre o quattro anni che viaggia liberamente sul

anche dalla scuola. Da lì formiamo i cittadini di domani e sarebbe davvero importante infondere a scuola anche questi principi che ci salvano davvero la vita, e non è un eufemismo.

approfondimenti ed esperienze su queste tematiche. Anche questi aspetti quindi potrebbero aiutare a ridurre le morti sul lavoro, perché si creerebbero *pool* di esperti per valutare i dati valutare i dati e le reali cause degli incidenti, potendo così fornire informazioni e supporti fondamentali, per fare in modo che si riducano finalmente e sul serio queste morti ingiuste. Mi auguro quindi che la mozione che oggi stiamo discutendo costituisca il motore e l'impulso per far sì che il Parlamento, in questa legislatura, vari provvedimenti che non sono più procrastinabili.

partire da questo dato numerico, che rappresenta il numero dei morti sul lavoro da gennaio a luglio 2023. È una fotografia relativa ai dati di quest'anno, che ci restituisce l'INAIL e che definirei raccapricciante. In Italia si continua a morire di lavoro, con dimensioni e una frequenza che non possiamo più tollerare e l'ultimo terribile incidente - che oggi ultimo più non è - che ci ha portato a discutere in quest'Aula, accelerando un processo che era comunque avviato, è quello di Brandizzo, in cui hanno perso la vita cinque persone. Dietro questi morti c'è il dramma di intere famiglie, che improvvisamente perdono i loro cari senza potersene fare una ragione, spesso purtroppo anche con la consapevolezza che quella perdita si sarebbe potuta evitare. Salutano i loro congiunti quando escono di casa per quella che dovrebbe essere una routinaria giornata di lavoro, ma poi non li vedono più tornare. Ovviamente in tutto questo c'è la responsabilità di tanti, innanzitutto dei datori di lavoro, che spesso si sottraggono al rispetto delle normative, nonostante siano obbligati a osservarle per garantire ai lavoratori la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.

ancora, chiaramente la responsabilità di noi politici e amministratori chiamati a legiferare e amministrare la cosa pubblica con la massima attenzione e lungimiranza possibile, ponendoci in questo caso come obiettivo l'abbattimento dell'incidenza degli infortuni, agendo su più fronti (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione e incentivazione), cosa che purtroppo fino a ora non è stata fatta. Nonostante in Italia abbiamo un impianto normativo definito dallo stesso ministro Calderone qualche giorno fa molto corposo, chi ci ha preceduto non è riuscito a far nulla di concreto perché quell'impianto desse i frutti attesi, evitando dunque i numerosissimi incidenti che si sono susseguiti.

il ministro Salvini con estrema contrizione ha ribadito che non si può morire di notte sul lavoro per errore umano e per mancanza di comunicazione e che bisogna garantire la sicurezza ai lavoratori sui cantieri e questo diventa più che mai urgente e necessario. Conoscendo la sua fortissima attenzione al tema al tema della sicurezza in generale, siamo certi che la questione non passerà senza interventi concreti. Suggeriamo, ancora, l'implementazione del fascicolo elettronico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'individuazione l'individuazione di *best practice* in materia, l'indicazione di nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento dei dati in forte sinergia con l'INAIL uno studio dell'eventuale relazione causale tra gli infortuni e la subfornitura o il subappalto di servizi. Anche questo argomento è particolarmente importante in questo momento in cui, grazie all'azione del Governo e *in primis* dello stesso ministro Salvini, che ha voluto e varato il nuovo codice degli appalti, diamo un nuovo impulso, per esempio, al settore dell'edilizia, nel quale subappalti e subforniture sono molto utilizzati e, piuttosto che bloccare i lavori, come sottolineo la necessità di intervenire sulla correlata questione della sicurezza sul lavoro. dell'opportunità di introdurre disposizioni di carattere premiale per le imprese che assicurano tutele maggiori, con la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e, al contrario, l'implementazione di misure disincentivanti per quelle che invece si rendano responsabili di violazioni in materia di sicurezza. Riteniamo che questo meccanismo possa essere utile per incidere sull'aspetto basilare della cultura della sicurezza e del cambio di mentalità Siamo tutti d'accordo poi sulla necessità di essere più presenti sulla formazione continua e sull'informazione, nonché sul parlare maggiormente di sicurezza anche nelle scuole, perché - appunto - è questione di cultura, di sensibilità e di prevenzione.

si può andare incontro ad incidenti spesso mortali, e dimostrando appunto come questa sensibilità e la consapevolezza in materia di sicurezza siano molto basse. Sensibilizzare ed educare a questo tema sono probabilmente le chiavi per riuscire davvero a ridurre gli incidenti e la base indispensabile da cui partire. Qualunque normativa infatti, per quanto eccellente possa essere, non è efficace, se non viene rispettata. E affinché sia rispettata, spesso non basta la sanzione per la sua mancata ma è necessario che sia introiettata, compresa, metabolizzata, fatta propria e accettata come giusta. Probabilmente, solo così le procedure da essa stabilite possono essere vissute ed applicate come normali. Concludo sottolineando anche come un ambiente di lavoro sano e sicuro, che garantisca al lavoratore un benessere psichico e fisico, influisca positivamente anche sulla produttività. È importante dunque agire anche su una cultura della sicurezza, oltre che sulle regole, guardando la questione anche da quest'angolazione. Questo è il nostro compito principale, ciò di cui ci stiamo occupando e su cui chiediamo al Governo di impegnarsi, cosa che sta già facendo e che continuerà certamente a fare, finalmente con una vera inversione di rotta rispetto al passato.

Signor Presidente, è doloroso e forse anche un po' frustrante dover constatare che anche questo pomeriggio i fatti, nella loro crudezza, hanno corso più veloce di noi. La seduta di oggi si svolge, ancora una volta, in una giornata di lutto per le vittime di Chieti, già ricordate dai colleghi e alle cui famiglie va ovviamente tutta la nostra vicinanza. Anche questo pomeriggio siamo arrivati troppo tardi. Questo succede proprio all'indomani del monito, già ricordato da altri colleghi, del presidente Mattarella, attraverso una lettera indirizzata alla ministra Calderone, che saluto e ringrazio per essere qui, come ovviamente saluto e ringrazio il ministro Salvini e il sottosegretario Durigon. Il presidente Mattarella, in modo inusuale, ha indirizzato una lettera alla Ministra del lavoro, in occasione di un momento di formazione per 800 ispettori del lavoro, il cui concorso è stato bandito tempo fa, già durante la scorsa legislatura, e ai quali noi speriamo si aggiungano presto nuovi colleghi, così ponendo rimedio allo storico sottodimensionamento degli enti preposti ai controlli, che è stato già richiamato. Il presidente Mattarella ha scritto che i morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza e che la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali e i luoghi di lavoro. di lavoro. L'avvio dei lavori della Commissione presieduta dal senatore Magni ci offre l'occasione di dimostrarci appunto permeabili, come il presidente Mattarella ci chiede, pronti di fronte all'urgenza di fare più e meglio. Il dubbio che questa seduta non si sarebbe tenuta senza la tragedia di Brandizzo si fonda purtroppo sulla considerazione che di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al di fuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, si discute ad intermittenza e solo quando la realtà ci dimostra, con la sua crudezza e violenza, quanto ancora ci sia da fare. fare. Gli incidenti e i decessi sul lavoro non sono e non possono essere considerati un dato fisiologico dell'attività produttiva o, peggio ancora, un suo effetto collaterale, ma sono sempre frutto - - o della disapplicazione delle norme o di mancati investimenti o di eccessiva compressione dei tempi e dei costi dell'organizzazione produttiva o comunque di altre variabili, su cui è possibile intervenire, con buone norme, con i controlli e con la cultura della prevenzione già richiamata. Io voglio ringraziare il presidente Magni in termini non rituali, perché ci ha condotti ad affrontare la discussione di oggi sulla scorta di un documento unitario della Commissione che, accantonando le divisioni politiche, pone le giuste domande e richiede al Governo impegni concreti e realizzabili. Voglio credere

Della mozione non dirò molto, ma voglio richiamare solo tre punti, poiché altri colleghi ne hanno già richiamati altri. Il primo: il faro che la mozione accende sulla catena di appalti e di subappalti, con lo scopo di indagare quanto e se la frammentazione organizzativa del ciclo produttivo incida sulla sicurezza per ragioni organizzative, di compressione di tempi, di costi e di controlli, al di fuori dell'accettabile, dell'accettabile, ma anche per la mancata consapevolezza da parte dei lavoratori dell'intero ciclo produttivo. Sappiamo che maggiore è il controllo, ossia la consapevolezza della propria mansione all'interno del ciclo, e minori sono i rischi e i pericoli. Il codice degli appalti, che è stato recentemente riformato, non sembra farsi carico a sufficienza di questi aspetti, molto concedendo alla compressione dei costi e alla deroga da precedenti discipline.

non possiamo permetterci che il Piano di ripresa e resilienza non sia massimamente attento alle condizioni di lavoro, avendo tra i suoi scopi proprio il sostegno all'occupazione e non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Dovremmo poi indagare meglio l'impatto delle nuove tecnologie, in termini di rischi e opportunità, sull'organizzazione e le condizioni di lavoro. Dobbiamo esigere che la tecnologia sia messa al servizio del miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, affinché il lavoro non diventi variabile dipendente di un calcolo algoritmico. Questo si fa attraverso la conoscenza e anche la regolazione. L'avanzamento tecnologico ci consegna algoritmi in grado di organizzare tempi e ritmi di lavoro in funzione della massimizzazione dei risultati e giustamente dei profitti, raramente però massimizzando la sicurezza e il benessere delle persone nel lavoro. Pensiamo a quello che succede ai *rider* - chi non ha visto sfrecciare nelle strade delle nostre città dei ciclofattorini? - o agli addetti alla logistica in termini generali, che sfrecciano e lavorano inseguendo gli ordini che un'intelligenza artificiale confeziona per loro. Un gran numero di questi lavoratori è rimasto vittima di infortuni anche gravi ed è per questo che l'Unione europea ci ha chiesto di agire affinché le aziende e le imprese rendano trasparenti gli algoritmi

il Governo abbia cancellato la norma che era stata introdotta dal ministro Orlando, durante la scorsa legislatura, con il Governo Draghi, che rendeva obbligatorio, in ottemperanza di una direttiva europea, rendere trasparenti questi algoritmi ai lavoratori e ai cittadini. Probabilmente la Commissione presieduta dal presidente Magni fornirà uno stimolo per fare ancora di più e ancora meglio, in ottemperanza di quella che - lo ripeto - è anche un'indicazione dell'Unione europea. L'ultimo e cruciale punto sul quale non mi soffermo, perché è già stato ampiamente trattato, è la rilevanza della cultura della prevenzione e delle *best* *practice.* Siamo in un Paese in cui, accanto a tante tragedie, è possibile enumerare anche tanti buoni esempi settoriali, aziendali e anche territoriali. Non lo farò qui, lo faremo in Commissione, ma ne cito solo uno perché mi ha visto in qualche modo protagonista e partecipe: nel 2015, in avvicinamento a quello che fu per la città da cui provengo, Milano, un grande evento, ossia l'Expo - probabilmente il ministro Salvini lo ricorda di tutela della salute (ATS), l'azienda sanitaria del territorio, la direzione territoriale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni datoriali e sindacali diedero vita al centro per la cultura della prevenzione sui luoghi di vita e sui luoghi di lavoro. L'obiettivo era far sì che quel grande evento, frutto dello sforzo di tutto il Paese e non solo di quel territorio, fosse a impatto zero dal punto di vista degli infortuni e delle morti sul lavoro. Quell'attività corale centrò l'obiettivo: in effetti, è possibile costruire opere ed eventi senza dispendio di vite e di sangue. È un piccolo esempio, segno di una collaborazione possibile e della non ineluttabilità della strage a cui assistiamo. Mi piacerebbe - e sono convinta che sia l'auspicio di tutti i colleghi - che questa Commissione, che oggi muove il suo primo passo, purtroppo ancora in un giorno di lutto, possa essere dimostrazione della capacità di protagonismo del Parlamento e di tutti noi in accordo con il Governo, sollecitandolo affinché le Istituzioni si rendano utili ai cittadini e ai lavoratori in difesa della dignità della vita e delle persone che lavorano. Auguro quindi a tutti noi un buon percorso.

la mozione unitaria discussa oggi in quest'Aula evidenzia quanto per tutti noi, per il Senato, sia una priorità assoluta il tema del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa mozione ha sicuramente un obiettivo ambizioso con l'introduzione, la revisione e il potenziamento di tutti gli atti finalizzati all'azzeramento degli infortuni e dev'essere conseguita attraverso un continuo, serio e costruttivo confronto. È necessario fare di più, senza dividersi e senza speculazioni politiche, uniti in questo intento.

di lavoro e soprattutto un approccio diverso alla gestione di tali rischi. Questo cambio culturale va però fatto da parte di tutti gli attori protagonisti: da una parte, dai datori di lavoro;

È necessario quindi dar vita a un processo di sensibilizzazione socioculturale, partendo da tutti i livelli di istruzione. Attraverso l'insegnamento nelle scuole, i ragazzi devono comprendere l'importanza della sicurezza sul lavoro, perché la vita potrà dire anche quando ci si sente invincibili. Questo percorso deve però essere costante, per far sì che l'esperienza che ci accompagna quando diventiamo più maturi non prevalga sull'attenzione e non si abbassi mai l'asticella

in maniera pedissequa la formazione, gli infortuni e tutte le informazioni che possono agevolare i processi per la gestione della sicurezza, così da permettere l'adozione di misure non solo astratte e generali, ma adeguate alla storia lavorativa di ognuno di noi, di ogni singolo lavoratore, come un vestito fatto su misura. Contemporaneamente, è necessario potenziare l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale. Rivolgo veramente un ringraziamento agli ispettori che quotidianamente controllano tutte le attività per l'Italia, cercando soprattutto quella sacca di illegalità che oggi non siamo in grado né di conteggiare né di verificare e quindi neanche di debellare. procedere, quindi, alla condivisione della banca dati per favorire questa interoperabilità tra strutture in modo da valutare, se possibile e se effettivamente esistente, la relazione causale fra gli istituti di decentramento lavorativo quali subvettura e subappalto - non dimentichiamo il distacco - e l'eventuale minore attenzione alla sicurezza accompagnata dall'aumento degli infortuni. un'azione di contrasto con un rafforzamento dell'impianto sanzionatorio, ma contemporaneamente valorizzare, attraverso politiche premiali che non devono per forza essere economiche, tutti quei datori di lavoro che assicurano queste tutele aggiuntive rispetto alle previsioni di legge. Occorre effettuare un monitoraggio continuo dei rilievi infortunistici per individuare gli impatti delle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini della prevenzione generale e specialmente degli infortuni sul lavoro. Tutto questo con l'obiettivo di prevenire, affinché la prevenzione, ove possibile, confezionata su misura con riferimento all'età, all'esperienza e ai settori lavorativi, possa veramente diventare lo strumento per rendere il lavoro più sicuro. Un ringraziamento va al Governo e *in primis* al ministro Calderone che da subito ha istituito un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Questo è un lavoro collettivo che ci coinvolge tutti e che ci deve trovare sempre presenti.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la mozione unitaria che discutiamo oggi in quest'Aula credo assuma un significato particolare all'indomani dell'incidente di Brandizzo, che ha scosso tutti quanti noi e certamente ha provocato un grandissimo dolore alla famiglia delle vittime, cui va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Vicinanza

Nel rendere il mio parere, quindi, sento il dovere di fornire al Parlamento alcuni aggiornamenti relativi all'attività del Ministero del lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di aggiungervi alcune mie considerazioni. Mi viene molto difficile parlare in questo momento, avendo ascoltato i vostri interventi e certamente avendo bene in mente che cosa significa implementare un percorso di salute e di sicurezza sul lavoro nell'ambito di un'azienda, che coinvolga in modo fattivo e in modo responsabile tutti Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta, come abbiamo sottolineato in altre occasioni, una priorità per il Governo e per il Ministero che va certamente conseguita anche attraverso un continuo e serio confronto con le parti sociali. Negli interventi precedenti si ricordava l'istituzione del tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, connesso al tessuto produttivo odierno e adeguato ai cambiamenti demografici e digitali e ai processi di transizione verde e a garantire la maggiore diffusione della cultura della sicurezza già a partire dall'istruzione scolastica per preparare le future lavoratrici e i futuri lavoratori. La cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, collegata ai principi basilari del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, si fonda sostanzialmente sulla conoscenza e sull'accertamento dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di lavoro e sulla capacità di un soggetto di conoscere e gestire questi rischi. Su questo punto e soprattutto dopo aver analizzato nel dettaglio alcuni dati forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, sono convinta che vi sia l'urgenza di avviare un corale processo di sensibilizzazione culturale con lo scopo di rendere la sicurezza sul lavoro parte integrante del patrimonio civico di ogni cittadino in ogni fase della sua vita. Questo obiettivo potrà essere raggiunto solo partendo dall'istruzione. Ha ragione il senatore Magni quando richiama la necessità di individuare dei percorsi di formazione specifica nell'ambito delle scuole. Bisogna fare in modo che nelle scuole, sin dai primi anni di insegnamento e con tutti gli strumenti utili, i nostri ragazzi maturino una più ampia e solida consapevolezza non solo del rischio, ma anche e soprattutto del rispetto della vita, la propria e quella degli altri. È proprio per questo che il Governo segue con favorevole attenzione l'*iter* d'esame delle proposte di legge attualmente incardinate in Parlamento che prevedono l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole, lì dove si formano le coscienze dei nostri ragazzi, del diritto del lavoro e in particolare della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo accompagnato questa prima fase, caratterizzata da una puntuale ricognizione dello stato dell'arte, con una spinta notevole sul fronte dei controlli. È stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'innesto di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023 sono stati assunti dall'Ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare agli uffici territoriali del lavoro, per i quali proprio ieri è stato inaugurato un corso di 175 ore, all'interno del quale sarà anche trattata specificamente la vigilanza in ambito ferroviario. Il tema della qualificazione e della qualità

importantissima sulla quale faremo tutti gli sforzi e metteremo in campo tutte le risorse necessarie, anche chiedendo il potenziamento con un ulteriore contingente. Come si ricordava precedentemente, abbiamo provveduto anche a gestire la giusta rivendicazione della perequazione delle indennità del personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro e abbiamo anche fatto un ulteriore intervento sul fronte della riorganizzazione dell'Ispettorato nell'ambito del decreto-legge pubblica amministrazione-*bis*. Questo *focus* appare veramente appropriato se richiamiamo gli eventi accaduti nel Comune di Brandizzo, però - come si è detto - oggi dobbiamo fare riferimento a tutte quelle situazioni in cui si perde la vita per motivi di lavoro, in occasione di Riferisco all'Assemblea che, nel merito della normativa applicabile in ambito ferroviario, risulta ancora vigente la disciplina in materia di trasporto ferroviario che risale al che risale al 1974, la legge n. 191, il cui articolo 35 prevede appunto che la programmazione delle attività di vigilanza viene svolta dall'Ispettorato del lavoro congiuntamente con il personale delle Ferrovie per la prevenzione degli infortuni. Nell'ambito delle sue competenze l'Ispettorato nazionale del lavoro ha da sempre condotto vigilanza nei settori produttivi ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nel settore delle costruzioni, con l'obiettivo di contrastare l'allarmante fenomeno degli infortuni. A partire dall'inizio di questa settimana, d'intesa con il Ministero, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha avviato un'attività di vigilanza straordinaria, denominata operazione Safety First, volta a una diffusa e capillare attività di controllo in edilizia e nei cantieri avviati per la realizzazione di progetti di efficientamento e di manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali realizzate sulla rete ferroviaria e stradale. Sono stati previsti controlli specifici sui cantieri caratterizzati da una elevata complessità progettuale e difficoltà esecutiva, per cui sono richiesti tempi rapidi di realizzazione o completamento che incidono sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro. I primi dati che emergono dagli esiti delle operazioni ispettive descritte, che sono ancora in corso, ci danno un quadro preoccupante, che deve indurre tutti - e sottolineo proprio tutti - quelli che hanno o hanno avuto responsabilità legislative, di governo, di gestione, di controllo o amministrative in materia di sicurezza sul lavoro a sentirsi in prima persona destinatari del messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto, mio tramite (non è inusuale, ero il soggetto che ha letto il messaggio), agli ispettori del lavoro che si accingevano a iniziare la loro formazione tecnica. In questo messaggio il Presidente sottolinea che il nostro Paese colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica. Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro. La cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro. È proprio la diffusa disapplicazione delle norme che dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro che sembra emergere dalle prime risultanze dell'operazione di cui vi ho parlato. Nella sola giornata di lunedì 11 settembre sono stati mobilitati 600 ispettori, che hanno verificato 186 cantieri e ispezionato 382 aziende, rilevando delle disapplicazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'operazione è ancora in corso; daremo più ampi dettagli non appena sarà conclusa la prima fase e avremo la possibilità di avere un quadro generale della situazione. I controlli intensivi proseguiranno senza sosta e saranno sempre più approfonditi e sistematici nei prossimi mesi, così da fornirci una base dati completa e dettagliata, che metteremo a disposizione della Commissione di inchiesta. A questo proposito, desidero rivolgere il mio ringraziamento al personale ispettivo e alle Forze dell'ordine, che si trovano a operare molto spesso in contesti non affatto facili. A questa forte azione di contrasto si accompagnerà una decisa azione di adeguamento della normativa, con una particolare attenzione all'impianto sanzionatorio. Voglio ricordare che sul tema il Ministero del lavoro ha messo in atto già diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul piano delle tutele assicurative e per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023. È stato istituito un fondo per i familiari degli studenti che sono rimasti vittime di infortuni mortali in occasione di attività formative successivamente al 1° gennaio 2018. È stata estesa la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione a tutte le attività di insegnamento e apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Come si ricordava, è stato incrementato per l'anno 2023 il fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro. È stato ulteriormente elevato il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l'ampliamento dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, ora non più obbligatoria nei soli casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ma anche qualora sia richiesta dalla valutazione dei rischi. Sono state ampliate le tutele dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'utilizzo delle opere provvisionali che frequentemente sono causa di infortunio. È stato previsto un controllo e un sistema di controlli sui corsi di formazione per i lavoratori e le altre figure, al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dei falsi attestati. Tutto questo è sufficiente? Assolutamente no. I dati, seppure in diminuzione nel 2023 rispetto al 2019 (anno prima del Covid), ci dicono che che bisogna fare di più per garantire ai lavoratori le più ampie tutele in materia di sicurezza e per fare in modo che incidenti mortali e infortuni invalidanti al punto di compromettere le condizioni di vita di chi ne resta vittima non si verifichino più. Un ruolo strategico nella protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro è rivestito sicuramente dalla formazione, pertanto è preminente l'attività diretta a dare attuazione alla disposizione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tra le priorità del 2023

A questo riguardo è stato costituito un gruppo di lavoro istituzionale chiamato a predisporre una bozza di accordo da sottoporre alle parti sociali, al fine di assicurare il prosieguo dell'*iter* volto ad acquisire l'intesa in sede di Conferenza permanente per i Il testo è già stato trasmesso alle parti sociali, siamo in attesa delle osservazioni per poter poi completare in tempi brevissimi l'*iter* di approvazione. Si tratta di un accordo certamente più adeguato ai tempi e alle evoluzioni del mondo del lavoro, tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel corso della pandemia. È stata prevista e disciplinata la formazione del datore di lavoro, oggi divenuta obbligatoria. Ci tengo a sottolineare un aspetto. La formazione non è e non può essere percepita come un costo, così come non può essere percepito come un costo tutto ciò che richiede gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. non possono e non devono essere considerate solo dei formali adempimenti. Investire in formazione rappresenta, al contrario, il rafforzamento della consapevolezza che lavorare in luoghi sani e sicuri contribuisce a tutelare la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e dunque a contrastare il fenomeno degli infortuni. Gli impegni che tutti i Gruppi parlamentari propongono oggi al Governo rappresentano delle linee d'azione sulle quali ci sentiamo in dovere di dare riscontro e sui cui in alcuni casi, come ho detto in precedenza, stiamo già operando. È il caso del potenziamento del personale ispettivo e della condivisione delle banche dati per favorire l'interoperabilità tra strutture competenti.

dando la priorità all'attivazione di un'apposita sezione volta a realizzare lo scambio di informazioni in tempo reale tra INAIL, Ispettorato nazionale e sistema delle Regioni in tema di vigilanza e di sanzioni irrogate nell'ambito della medesima attività ispettiva sull'applicazione della legislazione inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il Ministero ha svolto un'importante attività di coordinamento nei rapporti tra INAIL e Regioni per l'accesso all'utilizzo, da parte di queste ultime a titolo gratuito, dei servizi SINP dei flussi informativi, del registro di esposizione e del cruscotto infortuni. Con ciò si intende garantire, alle strutture regionali e provinciali preposte all'attività di programmazione e pianificazione in materia di sicurezza, l'efficiente assolvimento delle finalità istituzionali e degli obblighi di legge. Avvieremo ogni collaborazione istituzionale necessaria a studiare gli impatti delle nuove tecnologie sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, per individuare i migliori e più innovativi strumenti a supporto delle normali pratiche di prevenzione, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti del Ministero e degli altri soggetti istituzionali coinvolti. Anche alla luce delle risultanze ispettive, è necessario definire la proposta relativa alla qualificazione delle imprese rispetto alla sicurezza dei lavoratori, nell'ambito di una più generale e strutturata ipotesi di meccanismi premiali rivolti alle aziende virtuose. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è al lavoro e continuerà ad assicurare la più ampia disponibilità a proseguire nella predisposizione dei provvedimenti previsti per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È un lavoro collettivo che investe tutti noi, dal Governo al Parlamento, passando per le sigle di rappresentanza delle parti coinvolte. È con lo spirito di massima collaborazione che accolgo con grande favore la mozione odierna e, con l'auspicio che il tema della sicurezza dei lavoratori possa uscire dal novero degli argomenti oggetto di polemica politica, esprimo, sull'intero testo, il parere favorevole del Governo e mi sento impegnata a riferire puntualmente all'Assemblea gli sviluppi delle attività sui vari punti e a collaborare con la Commissione di inchiesta.

che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e sul piano morale e che il diritto alla vita, alla salute e alla dignità del lavoro rientri tra i diritti inviolabili della persona. Anche il riferimento contenuto nell'articolo 1, che - ricordiamolo - al tempo della Costituente fu un alto compromesso, diciamo così, tra le culture politiche democratiche, è in qualche modo indicativo di una scelta politica molto precisa che si volle fare. Ci fu una lunga discussione all'interno dell'Assemblea costituente, quando si decise poi di scrivere la frase

fecero la Costituzione italiana, su questo punto specifico avevano degli elementi di dissenso e di divergenza. Ci fu un emendamento delle sinistre, mi pare a prima firma Togliatti, che chiedeva che la Repubblica fosse la Repubblica dei lavoratori, in qualche modo sul modello di quello che accadeva in altri Paesi dell'Est Europa. C'era invece un'idea portata avanti in particolare dal pensiero più liberale, di far riferimento non al lavoro, ma alla cittadinanza. Alla fine ci fu un emendamento, mi pare a prima firma di Amintore Fanfani, in cui per l'appunto fu costruito questo alto compromesso e si fece riferimento a quello che poi leggiamo oggi, scolpito nella Costituzione, cioè la Repubblica

cioè il diritto di ciascuno di noi, di ciascuna persona, a lavorare e, per l'appunto, a realizzarsi attraverso il lavoro. Il lavoro veniva inteso con quella dizione esattamente come un soggetto politico attivo, per così dire, un soggetto politico includente, capace di diventare una vera e propria pietra angolare della democrazia che stava nascendo.

molti giorni, perché si fece fatica a trovare una sintesi invece poi così straordinaria) perché penso che dobbiamo tristemente riconoscere che l'auspicio e la formula dei Padri costituenti davvero stridano in maniera drammatica con la condizione attuale del Paese. Credo che anche su questo si debba fare tra di noi un'operazione di onestà intellettuale e riconoscere che il tema della condizione del lavoro e dei lavoratori non è un problema soltanto italiano, ma mondiale.

due milioni di morti all'anno, più di qualunque altra guerra. Evidentemente l'Occidente, l'Europa e l'Italia non sono altro rispetto a questo dato, che quindi non riguarda soltanto quei Paesi in cui è ancora più sofferente e faticosa la condizione sociale dei lavoratori, ma pienamente anche il nostro Paese. Sono stati ricordati anche stasera i numeri drammatici; è stato ricordato come dietro a ogni freddo numero

che non stiamo facendo abbastanza; la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro» perché, ha sottolineato il presidente, «le morti sul lavoro feriscono il nostro animo, feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza». È evidente che si tratta di un appello che dobbiamo fare nostro con un impegno rinnovato a intervenire sulla materia del lavoro. Crediamo che anche la frammentazione del mondo del lavoro, il cambiamento gigantesco dell'organizzazione del lavoro e la precarizzazione siano essi stessi causa delle morti e degli infortuni. Riteniamo che la sicurezza, la prevenzione e la formazione vengano troppo spesso considerate soltanto dei meri costi sui quali risparmiare, mentre la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere l'assoluta priorità.

significativo e che sia un passo avanti importante. Si tratta dal nostro punto di vista di un testo certamente condivisibile: anche questo naturalmente è frutto di una sintesi, come ovviamente è in casi come questo, ma io penso che si tratti di una sintesi giusta e positiva. Penso anche che si possa lavorare nel corso delle settimane che verranno con revisioni, miglioramenti e affinamenti che si riterranno necessari, tenendo ovviamente fermo l'obiettivo dell'abbattimento degli incidenti sul lavoro da realizzare attraverso attività sinergiche, cercando di attivare tutti gli strumenti disponibili: la prevenzione, la vigilanza, l'assistenza, anche la repressione, l'incentivazione delle buone pratiche preventive, fino - come è stato detto da diversi colleghi e io sono d'accordo - all'emarginazione di quelle aziende che reiteratamente violino le forme previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza, cercando al contrario di valorizzare il più possibile le imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro. Parliamo anche del potenziamento degli organici, della professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza, della opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria, per esempio, nella categoria dei lavori usuranti, di misure premiali per quelle imprese che assicurano più tutele e più salde per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di sanzioni per le imprese che si rendano responsabili di violazioni in tema di sicurezza. Parliamo anche di un altro tema. Ha parole, allorquando fa riferimento ad un altro tema molto serio, quello della trasparenza degli algoritmi. Parliamo, evidentemente, di un complesso di questioni, non ultima anche la necessità che la cultura della sicurezza del lavoro sia promossa in riferimento ad ogni livello di istruzione e di formazione, al pari anche di un monitoraggio più stringente sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, anche rafforzando le tecniche e gli istituti di prevenzione, per adeguare gli interventi correttivi alla tipologia di infortunio. Non è

su un tema secondo me particolarmente significativo come quello della alternanza scuola lavoro. A mio avviso, non bastano semplicemente gli indennizzi. Naturalmente sono meglio di niente, ma ovviamente non bastano. Noi dobbiamo parlarne molto seriamente, perché sono state troppe le storture con le quali abbiamo avuto a che fare in questi anni. Naturalmente, annuncio il voto favorevole alla mozione anche da parte del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra.

Era una presa di coscienza, una pratica sociale che fino a quel momento era stata sconosciuta, ma era anche l'idea che la morte e gli incidenti non potessero essere meri effetti collaterali del profitto. Io ritengo che si debba partire da queste parole, perché penso che, oggi come allora, la salute non si vende. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, le morti sul lavoro non sono una tragica fatalità. Esse sono lo specchio di un mondo del lavoro dove, nonostante l'indubbia presa di coscienza da parte dei dei datori di lavoro e dei lavoratori del tema della sicurezza che c'è stata in questi ultimi decenni, persistono purtroppo ancora troppe forme di sfruttamento, alle quali se ne aggiungono sempre di nuove. Pensiamo ai lavoratori della *gig economy*, alle enormi condizioni di stress in cui vengono sottoposti da quelle *app*, che svolgono oggi una vera e propria funzione di caporali digitali e che sono alla base dei troppi incidenti di cui i fattorini, che attraversano sfrecciando le nostre città, sono spesso vittime. Pensiamo anche alle cooperative spurie nella logistica e nell'edilizia, che nascono soltanto per gestire una commessa o un subappalto. soggetti che si muovono tutti in ambiti dove la concorrenza è feroce e spesso sleale, dove l'affannosa ricerca della riduzione dei costi è attuata a svantaggio della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Pensiamo all'agricoltura, un settore nel quale, soprattutto in alcune Regioni, si registrano ancora forme di sfruttamento di una manodopera straniera e illegale, pagata pochi euro al giorno, con l'odioso fenomeno del caporalato e delle organizzazioni criminali che taglieggiano gli sfruttati. È in questi contesti, nei quali la dignità dei lavoratori non ha alcuna tutela, negli anelli più deboli e spesso invisibili di importanti filiere produttive, che si registra il maggior numero di incidenti e di morti. Infortunarsi sul lavoro, spesso con esiti mortali, oltre ad essere inaccettabile per il rispetto e la cura che si deve ad ogni vita umana provoca ripercussioni anche in ambito economico: l'INAIL ci dice che il danno economico causato da infortuni e malattie professionali condiziona circa il 3 per cento del PIL. Dunque, far capire al nostro sistema produttivo che il rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro sono benefici anche dal punto di vista economico, oltre che da quello etico, è essenziale per contrastare il fenomeno delle morti e degli incidenti sul lavoro. A tale riguardo, è particolarmente importante l'impegno n. 10 chiesto al Governo promuovere la cultura della sicurezza. È infatti con la cultura che si fa crescere anche in quest'ambito la nostra comunità; con la cultura e non con gli slogan, né con l'inasprimento delle sanzioni. Bisogna investire nella prevenzione che genera risparmi e premi, non nella repressione, che genera costi e sanzioni. Allo stesso modo, è importante per noi evitare norme che, in nome della velocità o del profitto, chiudano gli occhi sui controlli o determinino un mondo del lavoro dove lo sfruttamento è la regola. Sicurezza e lotta allo sfruttamento sono due facce della stessa medaglia. Votiamo convintamente a favore di questa mozione, come Gruppo per le Autonomie. Signor Presidente, «verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dalla mattina alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo»: c'è una assonanza triste tra i tragici fatti di Brandizzo e questi versi di un letterato peraltro della stessa terra piemontese, Cesare Pavese. Il volto, lo sguardo. Signora Ministra, colleghi, penso che tutti noi faremo fatica e non dovremo dimenticare lo sguardo di Kevin Laganà in quel video recuperato su Instagram. un video agghiacciante: «Se vi dico "treno", vi spostate dall'altra parte». È uno sguardo che ci interroga, che ci responsabilizza, che ci pone delle domande. Penso che noi, rievocando il senso etimologico di quella poesia, dobbiamo evitare che la nostra rischi di essere una parola inutile, un grido strozzato o, peggio ancora di fronte a questi casi, un'abitudine irrazionale, alla quale non possiamo e non dobbiamo arrenderci.

a quel lungo e quotidiano stillicidio, lungo tutta la Penisola, che anche oggi, come è stato ricordato, si è manifestato e concretizzato in mezzo a noi; e se vogliamo andare al di là della retorica, delle frasi di circostanza, delle parole di cordoglio, dei momenti di solidarietà che sono pure dovuti, ma che ci impongono di riuscire a fare un salto in più nella nostra veste e nella nostra funzione, dobbiamo innanzitutto domandarci cosa può e cosa deve fare la politica. c'è anzitutto una esigenza di fondo: noi dobbiamo sottrarre questo tema da un meccanismo che ormai è stantio, ripetitivo - mi verrebbe da dire logorroico - che pretende la nostra divisione manichea su ogni argomento che la cronaca o la storia ci sottopongono. insomma una politica che sappia elevarsi dalle meschinità e dalle piccinerie per affrontare, da una parte, con oggettività e, dall'altra, nel merito le questioni per elaborare le soluzioni. La nostra opinione è che lo sforzo unitario di oggi, che va salutato positivamente e per il quale ringraziamo tutte le persone e tutti i colleghi che si sono impegnati in uno sforzo di individuazione di un punto di caduta comune, va in questa direzione. È con questo spirito che vanno esplorate le tre vie di lavoro che ci aspettano: anzitutto - come ha ricordato anche la signora Ministra nella sua allocuzione - la via legislativa, relativa alla legislazione di settore in materia di sicurezza. Se c'è da riformare - e c'è da riformare - lo si faccia presto e bene. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in termini propositivi, emendativi e di approvazione se il testo sarà come deve essere. C'è poi una seconda questione che non va sottaciuta nell'esigenza del recupero non ai fini polemici, ma ai fini oggettivi dello spirito a cui facevo riferimento in precedenza. Essa è relativa a un'analisi sulla legislazione che sottende in particolare il tema

è quindi con spirito polemico, ma con atto di constatazione, che dobbiamo considerare che l'incrocio fra le assegnazioni senza gara, l'elevazione dei livelli per i quali si può evitare il meccanismo della selezione competitiva e l'allungamento della filiera dei subappalti costituiscono un elemento pernicioso. genera infatti una situazione che è fatta da una frammentazione, da una costellazione di piccole imprese che - come ci dicono i dati - sono quelle in cui è maggiore l'incidenza degli infortuni. E questa frammentazione porta alla difficoltà dei controlli, alla creazione di lavoratori precari e, in alcuni casi, anche a una facilità di permeabilità di infiltrazioni. Non basta però solo fermarsi alla riflessione di carattere critico, perché sarebbe fin troppo facile. Vogliamo fare una proposta, signora Ministro: perché non introduciamo - potrebbero magari cominciare a farlo le grandi stazioni appaltanti pubbliche,

che dimostrano di aver investito sul versante della sicurezza e che con la loro attività si esercitano meno infortuni? Dobbiamo andare nella strada della qualità e non della dequalificazione. La seconda strada, è quella della via amministrativa. È stato ricordato in questo contesto e in questo dibattito - e lo riprendiamo anche noi - il tema del potenziamento, della qualificazione e del rafforzamento della rete degli ispettorati del lavoro

la facile scorciatoia nella quale cadiamo come in una tentazione quasi invincibile di fronte ai casi di cronaca, che è quella tentazione della risposta panpenalistica *(Applausi)*, e cioè l'invenzione di un reato al quale affidare la maieutica della soluzione definitiva. Non è così. Queste cose funzionano se c'è uno Stato che funziona; se c'è un'articolazione della pubblica amministrazione che funziona, non se si utilizza lo strumento del codice penale pensando che quella sia la scorciatoia rispetto al fatto che non qualifichiamo e non rendiamo efficiente la nostra macchina della pubblica amministrazione e della magistratura.

ed è il concetto della persona come merce, un concetto che alberga in vari settori, in vari segmenti, in varie esperienze della nostra vita sociale di questo tempo. La persona è una merce a vari livelli; siamo merci nel momento in cui trasferiamo i nostri dati su *big data* che ci utilizzano, ci controllano e ci subornano; sono merci quelle ragazze che vengono utilizzate per partorire in maniera impropria e che usano il loro corpo per far utilizzare i bambini che poi vengono venduti *(Applausi)*; sono merci gli operai che vengono buttati senza alcuno scrupolo dentro una fornace senza controllo e senza garanzia. Il rischio è che, se non ritroviamo un'etica condivisa attorno al valore della persona, non ritroveremo il legame che ci unisce in quanto comunità *(Applausi)* e, quindi, non potremo rimarginare le ferite di questo tempo, perché da sole le soluzioni legislative e le soluzioni tecniche non bastano. È quindi dall'esito delle nostre scelte che dipenderà se in futuro per riprendere le parole di Cesare Pavese - scenderemo nel gorgo muti come stanno purtroppo scendendo le famiglie dei ragazzi di Brandizzo e tante altre famiglie colpite da questi drammatici eventi o se sapremo, come dobbiamo, dare un indirizzo di speranza a questo Paese.

La risposta a questa domanda, purtroppo, ce l'ha data ancora una volta la spietata cronaca delle ultime settimane e purtroppo anche di qualche ora fa. Gli incidenti sul lavoro vengono definiti "morti bianche", in verità di bianco c'è ben poco: davanti a noi abbiamo il rosso del sangue e il nero del lutto, come se a provocarli non ci fossero una o più mani omicide. I numeri sono impietosi nella loro freddezza, perché da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, con una media di 80 decessi al mese. Dietro questi numeri ci sono storie di vita interrotte, famiglie distrutte, con mamme, papà e figli che si sono alzati presto la mattina per andare a guadagnarsi il pane quotidiano e che non sono mai tornati a casa. Sono storie e circostanze che ci colpiscono come cittadini e come lavoratori, ma che ci richiamano alla nostra responsabilità di rappresentanti del popolo e di legislatori a dare una risposta pronta e decisa. Quando si indaga sulle cause viene citata spesso l'imprudenza o la fredda decisione di ignorare tutte le norme di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, mettendo a repentaglio la vita per un minimo vantaggio, sia esso denaro in più o Molto spesso un lavoratore che perde la vita è vittima di azioni irresponsabili da parte di coloro che avrebbero dovuto garantirgli sicurezza, retribuzione appropriata e un futuro sicuro. La proposta che oggi siamo chiamati a votare vuole illuminare la strada ancora una volta alla ricerca delle risposte e delle soluzioni, con l'obiettivo di affrontare e vincere questa sfida. Non è sufficiente ridurre i casi di mortalità: l'obiettivo deve essere il loro completo azzeramento. Ecco perché con spirito di condivisione, consapevoli della terribile attualità del problema, ci impegniamo oggi a riportare al centro dell'agenda politica il tema della dignità e della sicurezza sul lavoro. Ha un colore politico questa battaglia? No che non lo ha. Devono essere strumentalizzati gli incidenti sul lavoro? Per onestà intellettuale non dovrebbero, anche se purtroppo ancora oggi assistiamo a occupazioni di piazze per individuare responsabilità istituzionali. Questa strage silenziosa e rumorosa al tempo stesso non nasce con questo Governo: esiste da anni e da anni attende soluzioni politiche e non mi pare che nell'ultimo decennio chi oggi fa la morale non si sia seduto tra i banchi del Governo. Per questo la sicurezza dei lavoratori richiede un impegno unanime da parte di tutti: non può e non deve essere una questione di parte. Invece di scendere in piazza per puntare il dito con pregiudizio e faziosità come ha fatto la CGIL - in questo processo per ottenere più sicurezza e meno vittime, i sindacati dovrebbero lavorare fianco a fianco con noi, con la politica, con il Governo, insieme con le associazioni dei lavoratori e con le imprese stesse. *(Applausi)*. Tutti hanno un ruolo cruciale nel rappresentare gli interessi dei lavoratori e nell'assicurare che le loro condizioni siano adeguate, serie e sicure. Dobbiamo agire con determinazione: il primo passo da compiere sicuramente è il rafforzamento della normativa sulla sicurezza del lavoro; è fondamentale che le imprese siano vincolate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e siano soggette ad aspre penalità in caso di violazioni. Pertanto, l'intensificazione dei controlli è di vitale importanza. I sindacati richiedono un aumento del numero di ispettori sul lavoro e questo Governo sta rispondendo con misure concrete. ha annunciato l'ingresso di 983 nuovi ispettori tecnici, confermando un impegno nel potenziare gli sforzi di prevenzione. Un monitoraggio adeguato e costante nel rispetto del norme di sicurezza può fare la differenza; rappresenta un deterrente che, seppur non decisivo, può svolgere un ruolo significativo. Non possiamo permettere che le aziende senza scrupoli eludano le leggi e mettano in pericolo la vita dei lavoratori con impunità. Inoltre, è importante promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso l'istruzione e la formazione a livello sia aziendale che individuale; un investimento nelle competenze dei lavoratori assicurerà la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione sul posto di lavoro; una cultura che parta dalle istituzioni, che devono incentivare la sicurezza sul lavoro, premiando le aziende che rispettano alti standard di sicurezza, anche attraverso l'implementazione dei modelli 231 e penalizzando quelle che adottano pratiche illegali. Questo richiede un'intensa attività di prevenzione e di monitoraggio che deve essere fatta in collaborazione con l'INAIL. Da non trascurare è anche il tema della completa defiscalizzazione dei costi per garantire la sicurezza: si tratterebbe di un importante incentivo per l'attuale situazione delle imprese nel nostro Paese. Alla luce di quello che ho appena detto, era del tutto inutile cercare di individuare un colpevole politico, anche in una terribile tragedia come quella di Brandizzo, puntando l'indice contro appalti e subappalti. Non è questo il punto. Sono previsti dalla legge e garantiscono la realizzazione delle opere pubbliche. Non è quello il problema è piuttosto una questione di come questi lavori vengono svolti. Chi controlla il rispetto delle norme che, tra l'altro, già esistono? Chi controlla che le procedure adottate siano quelle giuste? È poi possibile che con le nuove tecnologie ci si affidi ancora esclusivamente a telefonate e fonogrammi? Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che, mentre noi parliamo in questo nostro dibattito, ci sono famiglie affrante per lutti che è giusto definire inaccettabili. A loro dobbiamo risposte e garanzie, perché il sacrificio dei loro cari non sia stato inutile; dobbiamo assistenza e supporto dal punto di vista emotivo, psicologico e anche finanziario; dobbiamo garantire un accesso alle consulenze e al sostegno, nonché a indennizzi che devono essere giusti e tempestivi. Non siamo così superficiali da pensare che questa piaga trovi una soluzione dall'oggi al domani, perché siamo chiamati a un impegno a medio e lungo termine. Non dimentichiamo mai che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e che il diritto a un lavoro vuol dire anche il diritto a poterlo svolgere in sicurezza, senza paura, con le spalle coperte dalle aziende e da uno Stato che protegge e non abbandona, che sostiene e controlla il rispetto delle norme, accompagnando tutti coloro che tornano a casa ogni sera. sera. Il futuro dei nostri cittadini, di chi ogni mattina esce per produrre e rendere migliore questo Paese, dipende da noi e noi dobbiamo essere all'altezza di questa responsabilità. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

ministro Calderone, onorevoli colleghi, mi onoro di far parte della Commissione d'inchiesta che oggi ha presentato questa importante mozione, che deriva da un lavoro di squadra; finalmente una politica senza bandiere, su un obiettivo comune comune per il bene dell'Italia e degli italiani, sicuramente un po' mossa dalle tragedie che hanno riempito le nostre cronache. Ha sconvolto tutti quella di Brandizzo, che sembra inspiegabile; per i comuni cittadini sembra davvero inspiegabile. Purtroppo però, per chi vive quell'attività e quel lavoro, in maniera incredibile conferma che sono situazioni e tragedie purtroppo possibili. Questo ancor di più rende davvero increduli tutti noi, che siamo qui a rappresentare i cittadini e, quindi, il nostro dovere primario è occuparci di quanto è necessario mettere in campo per la difesa dei diritti. Il diritto al lavoro è uno dei diritti primari, a cui tutti dobbiamo dar seguito. Ho ascoltato con interesse tutti gli interventi e sono stata colpita da quello della ministra Calderone, che ha abbracciato

che spero davvero porti a un risultato utile per tanti giovani e cittadini che perdono la vita. I dati dell'INAIL confermano le gravi perdite, con numeri sempre in crescita. La cosa che colpisce è che anche i

fra gli *under* venti. Per contrastare la piaga degli incidenti non basta però la repressione, come abbiamo detto tutti. Le norme ci sono, ma nei fatti non vengono rispettate. Per prevenire è necessaria

necessaria una sinergia che deve abbracciare varie professionalità e varie posizioni sociali, professionali e politiche; la sinergia di tutto è necessaria. Purtroppo non sempre si investe in prevenzione e questo è confermato dagli incidenti che si verificano. Investire in prevenzione in prevenzione significa attenzionare gli strumenti messi in campo. Per questo nella mozione abbiamo parlato di premialità premialità per le imprese che investono in azioni utili alla prevenzione; una premialità che - come ha detto anche il presidente Magni, che ringrazio per il grande lavoro svolto

tutte queste azioni. Quindi, occorre una reale volontà per favorire il benessere dei propri collaboratori.

quindi essere messa a disposizione per evitare lungaggini. Non dimentichiamo che la semplificazione deve essere sempre un elemento imprescindibile affinché il tutto possa essere contestualizzato e concretizzato. L'incidente di Brandizzo pone sicuramente all'attenzione anche l'aspetto psichico e di fatica a cui possono essere sottoposti i lavoratori dopo tante ore di lavoro. Da qui la nostra proposta di inserire la manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti.

Nello stilare la lista di iniziative prioritarie ci sono dei punti ampiamente condivisi da tutti i Gruppi che hanno partecipato ai lavori della Commissione. Uno di questi è il riconoscimento del carattere culturale del tema della sicurezza, sicurezza, che deve rappresentare un tratto caratteristico di civiltà, quindi un elemento che dobbiamo perseguire proprio come tratto culturale di un'Italia civile, in un'impostazione che deve essere corale e collettiva.

renderci attivi anche rispetto alla volontà di rendere strutturale la formazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché la consapevolezza dei rischi è fondamentale. Per la prevenzione e la formazione nei luoghi di lavoro devono essere previste più risorse per incentivare i controlli.

essi ritengono di non essere numericamente supportati per poter affrontare la grande mole di lavoro. Forse anche questa forma di deterrente potrebbe essere utile a risolvere il problema, al fine di essere previdenti.

Signor Presidente, ministro Calderone, sottosegretario Durigon, colleghe senatrici e senatori, non si può morire di lavoro, non si può morire per lavoro, non si può uscire di casa e non tornare più per un incidente sul lavoro. La tragica morte dei cinque operai sui binari in un cantiere ferroviario di Brandizzo accende ancora una volta i riflettori sul dramma delle morti sul lavoro. Purtroppo, ogni giorno nel nostro Paese piangiamo perdite incomprensibili di vite umane, strappate alle loro famiglie e alle loro comunità. Non c'è solo il caso più recente: quello, purtroppo, è l'ultimo caso eclatante, ma ogni giorno ci sono almeno tre morti. Anzi, purtroppo, oggi abbiamo ricevuto dall'ANSA la notizia di un'esplosione in cui sono morti altri tre lavoratori. Dico "altri", perché in quell'azienda, addirittura recidiva, sono già capitati altri incidenti.

una grave perdita per tutti. È in gioco la dignità di noi stessi. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un frutto di tante responsabilità, economiche, sociali e anche politiche, che devono convergere sul servizio dei lavoratori. Come ha ricordato Papa Francesco, la sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno un valore inestimabile, agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore. Le tragedie più gravi, come quella di Brandizzo, squarciano il velo della disattenzione generale, polarizzano le attenzioni, ma dopo qualche tempo lo scandalo scema e la notizia, dalle prime pagine dei quotidiani, passa ai trafiletti, per poi sparire. Se andiamo ad analizzare gli esiti giudiziari, la sensazione è che queste morti siano avvolte da una dimensione di impotenza. I responsabili condannati devono scontare pene lievi, quasi simboliche. È successo ai dirigenti della multinazionale dell'acciaio ThyssenKrupp, responsabili, nel 2007, di un'altra grande tragedia, in cui sette operai furono uccisi da un'esplosione nello stabilimento di Torino; così come ad Stephan Schmidheiny, ultimo proprietario della Eternit, fabbrica che, fino a pochi anni fa, negli anni Novanta ha prodotto cemento amianto, un materiale tossico che ha causato la morte di molte persone. Non sono casi isolati: questi decessi sono non fenomeni naturali, ma la diretta conseguenza di una ben identificabile organizzazione del lavoro e del modo in cui il lavoro è oggi considerato all'interno della nostra società. Il primo articolo della Costituzione dice che «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro» e i nostri Padri costituenti consideravano il lavoro un elemento centrale della democrazia, non in senso astratto. una centralità che, fino alla seconda metà del Novecento, ha consentito di ottenere importanti conquiste, in termini non solo di remunerazione e condizioni lavorative, ma anche di *status*. Fare l'operaio era uno *status*, anzi, dava un lavoro, uno stipendio sicuro, una sicurezza per la famiglia e anche per il futuro, un lavoro che permetteva di pensare a costruire una famiglia, a comprare una casa, a programmare le vacanze o a fare altri investimenti. Oggi i lavoratori non hanno autorevolezza, non sono più considerati protagonisti della vita collettiva e non godono del riconoscimento. Il lavoro manuale ha subito un processo molto violento di marginalizzazione economica, sociale e culturale. I morti di Brandizzo facevano un lavoro manuale, quelli che svolgono compiti faticosi e pericolosi, ma retribuiti, e che riempiono le cronache con le loro morti, di cui ci si dimentica in fretta. Protagonisti della società sono invece imprenditori, finanzieri, ma soprattutto gli *influencer*, soprattutto quelli dalla vita e dai soldi facili. Da più di venti anni gli stipendi nel nostro Paese sono al palo. L'Italia è l'ultimo Stato dei Paesi dell'OSCE e l'unico in cui salari non si sono adeguati in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi. Abbiamo perso anche la dimensione di carriera: il lavoro consiste in impieghi di breve durata, non correlati tra loro, per cui non esiste più il percorso su cui costruire la propria vita ed è naturale che i giovani non ci vogliano investire. Altro punto importante è l'esternalizzazione dei servizi, degli appalti e dei subappalti, che sono pericolosi perché permettono di ridurre al minimo la responsabilità, che viene così distribuita tra una miriade di soggetti e rende più difficile la comunicazione interna. Al tempo stesso i ritmi diventano insostenibili; i contratti a termine sono un cappio al collo che obbliga a rispettare determinati tempi. Le esternalizzazioni e gli appalti usati anche da società pubbliche rivelano direttamente quella logica di massima efficienza, aumento dei profitti

È necessario quindi individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni, che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga contro, tra l'altro, del principio di differenziazione delle attività economiche e dell'evoluzione del mondo del lavoro. È necessario un più efficace ed efficiente coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla vigilanza sul lavoro. La riforma del sistema ispettivo realizzata a costo zero ha determinato una mancanza di investimenti in infrastrutture materiali, ma soprattutto di risorse per contrastare l'annoso problema del lavoro nero e irregolare, che porta con sé l'evasione fiscale e contributiva. Aggiungo anche che, oltre alla mancanza degli ispettori, bisognerebbe - a detta degli stessi che sono venuti in audizione alla Camera nella scorsa legislatura - semplificare le loro procedure e lasciarli più operativi sul campo e non chiusi negli uffici a compilare delle carte. Possono essere una risorsa importante per l'attività di formazione e preventiva per la sicurezza sul lavoro, così da non essere visti solo come controllori e sanzionatori. Gli appalti al massimo ribasso mettono sempre in secondo piano la sicurezza. All'epoca dell'intelligenza artificiale e di tecnologie sempre più evolute non ci possono essere errori di comunicazione: serve un sistema premiale per chi rispetta le regole e un sistema punitivo fino all'espulsione dagli appalti pubblici per quelle imprese che hanno comportamenti scorretti che provocano incidenti sul lavoro. È fondamentale predisporre subito più efficaci procedure e nuovi controlli per costringere le ditte a rispettare maggiore sicurezza. Non possiamo più consentire che si muoia sul lavoro per il mancato rispetto di norme di sicurezza basilari.

per l'attenzione a questa importante tematica e tutti i parlamentari che hanno firmato questa mozione unitaria e che voteranno naturalmente a favore. Sicuramente deve essere fatto un lavoro collaborativo

fare quadrato per portare a regime le attività espresse all'interno della mozione. L'impegno della Lega è in prima linea per tutti i lavoratori perché non si può morire di lavoro.

confesso che non riesco a non essere pervasa da una rabbia dopo le notizie che sono giunte oggi pomeriggio: non solo per la tragedia di altri operai che hanno lasciato la vita in un'esplosione in una fabbrica, ma perché, in realtà, se ripercorriamo la cronaca di quella stessa azienda, ritroviamo, poco tempo fa, un'altra strage, con le stesse caratteristiche e anche lo stesso numero di morti e, negli anni precedenti, degli altri infortuni mortali, sempre nella stessa azienda. La collega Tajani, intervenendo oggi pomeriggio, diceva che anche oggi siamo arrivati tardi. Credo sia assolutamente vero: parole che dovremmo scolpirci nella mente. Siamo di fronte a delle terribili contabilità, che però ci dicono che quegli eventi si ripetono e che non subentra un ragionamento, un pensiero, una domanda: se valga la pena; se sia possibile pensare che delle attività siano così profittevoli o interessanti da mettere nel conto la possibilità di avere ripetute morti di lavoratori e di lavoratrici.

sono i numeri, non di qualche fatalità, ma sono i numeri di una guerra, che continua a esercitarsi e che prosegue implacabile e ripetuta negli anni. Se noi guardiamo la sequenza storica dei numeri degli infortuni, quelli ufficiali, quelli registrati dall'INAIL, vediamo ben poche oscillazioni e vediamo anche che quei numeri si ripetono e che si ripetono le tipologie degli incidenti. Smettiamo di parlare di morti bianche, di fatalità, di tutto ciò che cerca di dare l'idea che questa sia una realtà impossibile da prevenire e che dobbiamo abituarci a subire. Invece, cominciamo a ragionare su qual è il prezzo a che cosa si paga un prezzo per cui si muore sul lavoro. Ragioniamo sul perché lavoratori e lavoratrici devono pagare questo tributo alla pressione del continuare ad aumentare i ritmi, alla pressione di fare di più e di fare più in fretta, a una visione miope che spesso ci ha portato a discutere dei temi della sicurezza in ragione di costi da evitare e non in ragione di investimenti per la difesa delle vite. noi stessi che non si può dire e non si può accettare che il profitto sia più importante di quella cosa essenziale che è tutelare la vita e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed è per questo che, se non entra nel nostro linguaggio l'abitudine a dire prevenzione sulla sicurezza, ma solo analisi *a posteriori*, difficilmente faremo dei grandi passi avanti. Così come forse dobbiamo cominciare ad avere l'abitudine di pensare non solo alla punta dell'*iceberg*, a quel drammatico numero di morti sul lavoro, anche a cosa succede ai tanti che subiscono infortuni magari non mortali, ma invalidanti; a cosa succede a quegli sconosciuti, di cui non parliamo, ma che contraggono sul lavoro malattie professionali gravissime, e di cui magari scopriamo le ragioni della morte anni e anni dopo. però ci interrogassimo tra noi, ognuno direbbe che la vita è la cosa più importante e che l'impegno di proteggere le vite è per noi un imperativo collettivo. Se è così, dobbiamo allora porci due questioni. Una la ponevo prima: dove sta l'asticella? A che punto cominciamo a dire che non vi è ragione possibile perché si mettano a rischio delle vite? questione, illustrata già dal collega Lombardo nel suo intervento, è l'universalità dell'assicurazione contro gli infortuni, la possibilità che chiunque lavori nel nostro Paese abbia la certezza di avere una copertura assicurativa. Se cominciassimo a ragionare in termini di prevenzione, probabilmente cambieremmo anche l'atteggiamento rispetto al tema dei costi, oltre al fatto che cominceremmo a considerare che le persone non sono mai l'equivalente del costo di una merce. Non lo possono essere proprio perché, innanzitutto, è la sicurezza, l'interazione diretta con i loro corpi, con le loro peculiarità, con la loro esistenza che non può essere messa in discussione.

e che quindi dobbiamo fare di più, perché sono i numeri di una guerra e non di una fatalità. Se gli infortuni si ripetono nelle loro modalità, questo ci permette di ragionare su come contrastarli su come contrastarli e sul fatto che i numeri che non conosciamo sono quelli che derivano dal sommerso, dalle irregolarità e dai caporali di quei lavoratori che magari vengono nascosti in un ciglio della strada perché non si sappia che c'è stato un incidente o di quelli che sono stati assunti poche ore prima dell'incidente. Sono Sono i numeri di modalità e di tecniche di lavoro che non investono sulla prevenzione e sulla sicurezza e che non usano la tecnologia. È sempre difficile parlare di una tragedia che è avvenuta, però una domanda possiamo farcela: perché nelle centrali di controllo ci sono visori che permettono di vedere chilometri e chilometri della ferrovia o di un'autostrada,

formula invisibile matematica che però detta le condizioni di lavoro alle persone, i turni e la velocità, ma ha anche la faccia degli strumenti che ci permettono di vedere, di prevenire e di dare modalità diverse di prevenire gli incidenti sul lavoro. Sta alla responsabilità politica, alla nostra responsabilità, decidere se la tecnologia la utilizziamo in una direzione o nell'altra. Se permettiamo che non ci sia trasparenza nell'uso degli algoritmi, in realtà abbiamo già scelto che la direzione è quella del mancato rispetto delle persone. Penso per esempio a un numero che non compare negli infortuni: i *rider* non sono assicurati, perché non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto all'assicurazione generale. *(Applausi)*. Questo vuol dire che o se la pagano loro o non hanno la possibilità di averla. E allora, quello è un uso della tecnologia, mentre un altro è dire che un sensore

Insieme - l'hanno detto tutti i colleghi e le colleghe - bisogna fare grande attività di formazione e di cultura, cominciare prima e determinare il fatto che sia normale affrontare il lavoro e prepararsi ad esso avendo formazione. Insieme però ci vogliono i controlli, perché quel mondo sommerso e quel mercato del lavoro deregolato che fanno tanta parte anche dei problemi della sicurezza hanno bisogno di controlli.

risorse e scelte perché gli ispettori siano di più. Con questa dichiarazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla mozione, ringraziando

sempre accesi, come sprone per quello che dobbiamo fare, perché - ci direbbe un cantautore - per quanto ci possiamo credere assolti - cosa che avviene ogni volta che si spengono le luci in realtà siamo tutti coinvolti e siamo lo stesso coinvolti. È esattamente per questo che il voto che questa Camera esprimerà rispetto alla Nazione dev'essere una scelta pubblica di coinvolgimento, un impegno e un dovere verso i lavoratori e le lavoratrici. Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, è vero, interveniamo in una giornata di lutto, ma se i numeri sono quelli che ci comunica l'INAIL, che purtroppo però non sono quelli, perché sono di più, facendo una divisione, ogni giorno c'è un lutto in Italia: che rabbia, che tristezza, che amarezza! Pensare che si esce la mattina di casa per andare a guadagnarsi un tozzo di pane e portarlo poi la sera alla famiglia e, invece, durante la giornata può succedere ciò che uno mai avrebbe immaginato: una tragedia. tragedia. Pensavo, sbagliando, che dinanzi a queste problematiche, a queste tragedie, ci fosse unione e non speculazione mediatica da parte di colleghi politici.

Non possiamo piangerci addosso, ci dobbiamo rimboccare le maniche e dare il nostro modesto contributo. Non sono d'accordo con quel collega che ha detto che non riusciamo ad incidere: io invece sì, io voglio incidere.

i ragazzi sono sacchi vuoti da riempire e noi dobbiamo riempirli. Noi dobbiamo inculcargli il concetto della cultura della sicurezza, perché purtroppo è quello che ci manca. Ve lo dice un addetto ai lavori. Quando avvio lavori in qualità di responsabile della sicurezza e faccio l'informazione ai lavoratori, vi posso garantire che cerco di terrorizzarli.

devono cercare di lavorare in sicurezza. Sono convinto di essere ascoltato, ma mi illudo, perché poi mi capita di vedere un lavoratore che, anziché utilizzare una scaletta per salire su un'impalcatura, si arrampica come una scimmia all'impalcatura stessa. Lì naturalmente parte la parte la rabbia e, in qualche modo, per quello che posso, intervengo. Ma con chi ce la vogliamo prendere, se un *influencer* sale su una gru alta 25 metri per farsi un video o un *selfie* da pubblicare su Tik Tok, e poi, purtroppo, cade e muore?

possiamo dare il nostro contributo per mettere mano al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, facendolo sulla scorta delle esperienze vissute e di ciò che purtroppo ci capita. Sono d'accordo: Sono d'accordo: una delle proposte che farò è proprio quella di istituire un documento tipo il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dà la possibilità alle imprese di partecipare alle gare e di lavorare solo se in regola con i contributi. Proporrò allora il DURS, visto che parliamo di acronimi, il documento unico di regolarità sulla sicurezza e dobbiamo studiare anche una sorta di premialità e di penalità, perché a un'azienda ligia al dovere, che fa lavorare i propri lavoratori con tutti i criteri sulla sicurezza, va riconosciuta una premialità, che può essere anche un privilegio, una sorta di prelazione nel momento in cui partecipa a una gara o a un bando di finanziamento indetto proprio dall'INAIL in materia di sicurezza sul lavoro. Allo stesso modo, è opportuno prevedere una penalità per le imprese e per le aziende che non fanno lavorare i propri lavoratori in sicurezza ed eventualmente arrivare anche a radiarle dall'elenco delle imprese e non farle lavorare, per vedere se poi effettivamente si adeguano o meno, perché la mia convinzione

- e quello che manca è un coordinamento fra di loro. Ve lo dico perché mi capita di avere cantieri dove nell'arco di un mese arrivano tutti gli enti e cantieri dove per sei o sette mesi invece non si vede assolutamente nessuno. Forse, allora, sarebbe opportuno pensare a un coordinamento tra tutti questi enti preposti, i quali possono calendarizzare e programmare sopralluoghi e visite ispettive, perché vi posso garantire che, quando circola la voce in una città che ci sono gli spettatori in giro, l'impresa che non è a norma sospende l'attività per quel giorno e cerca di adeguarsi, oppure c'è l'impresa furba che sospende, in attesa che vadano via i controlli e poi ritorna a lavorare. Allora, solo per il fatto che a cadenza quindicinale potrebbe arrivare un'ispezione, forse forse ci si penserebbe tre volte prima di mettersi a lavorare senza rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È una buona

applico e mi sono reso conto che funziona: come abbiamo il direttore di cantiere che controlla le lavorazioni, prevediamo il direttore di cantiere specializzato in sicurezza,

si può entrare solo quando si è in regola, quando si hanno tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale, quando si è a posto con la documentazione sull'assunzione

a controllare quello che effettivamente si fa. La sicurezza non è solo la redazione di un piano in materia, secondo il quale purtroppo - mi duole dirlo - spesso tanti colleghi fanno copia e incolla o probabilmente fotocopiano il documento (e questo, da professionista, non vi nascondo di averlo sempre contestato, ma non sono riuscito

Naturalmente, potremmo pensare di tutto e di più. perché l'obiettivo nostro è quello di dare un contributo per cercare di risolvere il problema e sono convinto che solo stando uniti lo si possa fare. Stasera è emersa una volontà unanime di stare uniti, perché effettivamente questo tema è così importante che dobbiamo necessariamente affrontarlo insieme. in qualità di rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, che mi onoro di rappresentare, esprimo il voto favorevole alla mozione

È naturale che sia così, per la portata di quell'attacco e di quella tragedia e per la risposta forte e unitaria che le forze e i Paesi democratici di tutto il mondo diedero a quell'offensiva del terrorismo. Per la mia generazione ci fu, cinquant'anni fa, un altro 11 settembre: quello in cui in Cile un colpo di Stato guidato dal generale Pinochet appoggiato di fatto dagli Stati Uniti pose fine all'esperienza democratica di Salvador Allende e alla stessa vita del presidente socialista al Palacio de la Moneda. Ci furono un'emozione e una commozione grandissime in tutto il mondo. In un'America Latina dominata da dittature fasciste e regimi militari, l'Unidad Popular di Allende aveva suscitato speranze e solidarietà: una vittoria democratica, un'esperienza di governo difficile, anche con errori, ma bella, accompagnata da quella musica andina, simbolo di libertà e creatività, come le poesie di Pablo Neruda. Era la prima esperienza delle sinistre al potere con le armi della democrazia: cinque anni prima, per la verità, c'era stato in Europa a Praga il tentativo di Alexander Dubcek, ma ci pensarono i carri armati sovietici a schiantare quel tentativo e il sacrificio di Jan Palach è ancora nella memoria collettiva. Il Cile di Allende segnò un'intera generazione. L'Italia e l'ambasciata italiana a Santiago si spesero più di tutti per dare sostegno a centinaia di antifascisti cileni, riusciti a fuggire dai massacri dello stadio di Santiago. Ricordo ancora con emozione il 18 novembre del 1973: eravamo più giovani, c'eravamo alla grande manifestazione di Piazza San Carlo a Torino, nella quale parlarono Isabel Allende, un delegato del consiglio di fabbrica della Fiat e il presidente della Camera Sandro Pertini. Ricordo i tanti cileni che vennero ospitati in Italia, in tante Regioni; ricordo nella mia Umbria l'emozione di avere gli Inti-Illimani, di avere Charo Cofré e *Hugo Arévalo*, di avere Juan Barattini, Marta Contreras. Pensate: Claudia Claudia Barattini, la figlia di Juan e Marta, decenni dopo, quando in Cile tornò la democrazia, divenne ministro della cultura di quel Paese. Presidente, ho finito: "Cile libero!", gridavamo alle assemblee scolastiche e alle manifestazioni, dove le bandiere rosse dei comunisti italiani e dei socialisti si confondevano con quelle democristiane, con quelle degli altri partiti democratici, con quelle dei sindacati, perché quel Cile e Salvador Allende furono davvero un simbolo di libertà per l'America Latina e per il mondo. È importantissimo aver visto condannati alcuni di quei militari, tra cui quelli che tagliarono le dita a Victor Jara, il cantautore, per impedirgli di suonare la chitarra, che poi uccisero con la terribile e crudele roulette russa. È È giusto, io credo, ricordare e rendere omaggio a quell'esperienza, cinquant'anni dopo, per non dimenticare il Cile di Allende e perché la democrazia e la libertà sono conquiste non definitive, da difendere e far vivere ogni giorno.

Signor Presidente, oggi è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge del Governo che reca «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazione alla circolazione stradale». Questo decreto-legge muove dalla necessità di dimostrare all'Unione europea l'impegno dell'Italia a rimuovere le ragioni per cui si trova sotto procedura di infrazione per il superamento sistematico e continuato delle soglie massime di emissioni nocive per la salute, come le polveri sottili, nelle Regioni del Nord Italia principalmente, che vede la Lombardia in prima fila. Questo decreto-legge sembra sottovalutare l'urgenza di intervenire per evitare la morte e la malattia dei cittadini a causa della pessima qualità dell'aria che respirano. L'inquinamento atmosferico continua a mietere vittime e le politiche per la qualità dell'aria falliscono per mancanza di una determinata volontà politica. Forse occorrerebbe riflettere meglio sul senso e sul valore delle prescrizioni europee e delle procedure di infrazione. Sono misure a tutela della vita e della salute dei cittadini, non sono fini a sé stesse, per infastidire i pendolari e gli utenti della strada. Questo decreto-legge mi lascia un po' perplessa, laddove al secondo comma dell'articolo 1, per esempio, prevede che le Regioni interessate dalla procedura di infrazione UE per il superamento delle soglie minime di emissioni di agenti inquinanti nocivi per la salute possano disporre la limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti solo ed esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Mi chiedo quindi, se qualche Regione virtuosa volesse pensare alla salvaguardia della salute dei cittadini in un momento precedente al 1° ottobre 2024, non potrebbe farlo? prosegue stabilendo che le limitazioni alla circolazione saranno inserite nei piani della qualità dell'aria regionali a decorrere dal 1° ottobre 2025; quindi, ancora due anni sotto infrazione e ancora morti per inquinamento, l'autonomia locale e l'autonomia decisionale vanno a farsi benedire. Mi chiedo se tra le priorità di questo Governo sia annoverata la tutela della salute e della vita dei cittadini. Quante morti dovremo ancora avere sulla coscienza, da oggi al 2025, prima di comprendere che la salute è più importante della possibilità di circolare liberamente e ovunque con un veicolo inquinante? Abbiamo appena pianto le morti sul lavoro oggi, ma non consideriamo che esistono morti altrettanto ingiuste causate dall'aria che respiriamo e che non riusciamo a migliorare. Secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), ogni anno, solo a causa delle polveri sottili PM 2,5, in tutto il Paese muoiono 60.000 persone in modo prematuro. Il *record* spetta alla Lombardia: sono 15.170 i decessi prematuri della Regione, 4.000 in tutta la città metropolitana di Milano. È una questione di priorità. Il non condivisibile ordine di priorità di questo Governo si manifesta anche parallelamente a livello regionale: mi riferisco alla Regione Lombardia, sotto procedura di infrazione, a guida Fontana, dove proprio in questi giorni la Lega ha presentato una mozione che invita la propria Giunta a sensibilizzare il sindaco della città di Milano a mitigare le misure di limitazione all'ingresso in area B veicoli inquinanti. Il Comune di Milano infatti ha pianificato da tempo le limitazioni, prevedendo una deroga di 50 ingressi per il biennio 2022-2023, che scendono a 25 per il 2023-2024. La Lega chiede che vengano mantenuti 50 ingressi anche per il prossimo periodo, motivando la propria richiesta con il danno economico che la limitazione della circolazione provoca a cittadini e imprese. In conclusione, si tratta di miopia e cecità al Governo: cosa è più importante, la vita o il portafoglio? A cosa serve il portafoglio pieno, se si perde la vita? Da oltre un decennio in Lombardia non si registrano miglioramenti per l'inquinamento da polveri sottili che, com'è scientificamente noto, rappresentano un grave problema sanitario. I dati confermano che ci troviamo davanti a un problema che va combattuto con celerità e strumenti adeguati, ma questo Governo pare negarlo. Le decisioni politiche hanno una responsabilità ben precisa: morti evitabili. Le misure antismog devono partire da una presa di coscienza del problema e vanno finanziate da Regione, Stato e Unione europea, perché non vi può essere salute dei cittadini senza salute del pianeta. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: senatore Francesco Silvestro; Vice Presidenti: senatore Bartolomeo Amidei e deputato Claudio Michele Stefanazzi; Segretari: deputata Rebecca Frassini e senatore Daniele Manca. La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Presidente: deputato Alberto Bagnai; Vice Presidenti: senatore

Dondi e deputato Virgilio Merola.